Poiché non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione sugli emendamenti al decreto-legge in materia di contrasto alla scarsità idrica, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

Il relatore, senatore Borghesi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi Signor Presidente, l'Assemblea è nuovamente chiamata all'esame, in terza lettura stanti le modifiche introdotte al testo dalla Camera dei deputati, del disegno di legge recante la ratifica dell'accordo sottoscritto nel dicembre 2020 tra l'Italia e la Confederazione svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, nonché del protocollo, firmato sempre nel dicembre 2020 dai due Paesi, di modifica della convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, risalente al 1976 e più volte modificata. Ricordo che il testo approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura lo scorso 1o febbraio è volto a ratificare un'intesa destinata a sostituire quella attualmente in vigore, che risale al 1974, al fine di migliorare il dispositivo di imposizione dei frontalieri e segnare una nuova tappa nelle relazioni fiscali tra l'Italia e la Svizzera. La modifica apportata dalla Camera dei deputati ha riguardato l'adozione di uno specifico emendamento, presentato dal Governo, in materia di telelavoro, che ha aggiunto l'articolo 12 al disegno di legge di ratifica, nonché l'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 sugli Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. finestra"). Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo qui per discutere un provvedimento di fondamentale importanza per migliaia di lavoratori transfrontalieri e per i territori di confine tra Italia e Svizzera. Per troppo tempo, questi lavoratori e queste aree hanno dovuto confrontarsi con un sistema giuridico e fiscale antiquato e inadeguato, che non solo rendeva difficile la vita quotidiana di tante persone, ma rappresentava anche un ostacolo allo sviluppo economico e alla cooperazione tra i due Paesi. Finalmente, grazie a questo disegno di legge, siamo in grado di apportare le necessarie modifiche e modernizzazioni a questo sistema. Ma cosa significa concretamente questo provvedimento per i lavoratori transfrontalieri e per i territori di confine? Innanzitutto, stabilisce un nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera che, oltre ad adeguarsi alle esigenze del XXI secolo, garantisce un trattamento più equo e corretto per tutti i lavoratori coinvolti. In particolare, si prevede un aumento delle franchigie da 7.500 a 10.000 euro, un aspetto fondamentale per garantire condizioni più favorevoli per i nuovi lavoratori transfrontalieri. Inoltre, il provvedimento assicura la stabilizzazione delle risorse finanziarie destinate ai Comuni di frontiera, pari a circa 89 milioni di euro, fondamentali per garantire la qualità dei servizi e delle opportunità offerte a imprese e famiglie residenti in questi territori. A tal proposito, è importante sottolineare l'istituzione di un fondo per lo sviluppo socio-economico e infrastrutturale, che partirà da una dotazione iniziale di 1,66 milioni di euro, per arrivare, nel 2045, a oltre 220 milioni di euro, destinati a promuovere lo sviluppo infrastrutturale e a colmare il *gap* tra le imprese locali e quelle di confine. Tuttavia, non possiamo ignorare una questione ancora irrisolta: il telelavoro. Nonostante gli impegni assunti dal ministro Giorgetti, questo tema rimane ancora in sospeso, mettendo in difficoltà l'organizzazione della vita di molte persone, in particolare donne. In una società che tende ancora a ripartire in modo iniquo le responsabilità familiari e domestiche, le donne si trovano spesso a dover bilanciare impegni lavorativi e compiti familiari, con un impatto negativo sulla loro carriera, sul loro benessere e sulla parità di genere nel mondo del lavoro. Il telelavoro non rappresenta quindi un'opportunità concreta per ridurre questo divario, favorendo una migliore partecipazione delle stesse al mercato del lavoro e una migliore conciliazione tra lavoro e vita privata? Il telelavoro è infatti sinonimo di flessibilità oraria e di possibilità di gestire in maniera più efficiente le proprie responsabilità familiari, rappresentando una grande opportunità, ma affinché il suo potenziale si traduca in benefici concreti è necessario un impegno collettivo e una visione lungimirante da parte di istituzioni, datori di lavoro e lavoratori. Come potremmo poi non considerare l'impatto ambientale? Viviamo in un'epoca in cui i cambiamenti climatici rappresentano una grave minaccia al nostro pianeta e alle generazioni future. In questo contesto il lavoro può offrire un contributo significativo alla riduzione delle emissioni di gas serra e al contenimento del riscaldamento globale. La diminuzione degli spostamenti quotidiani casa-lavoro contribuisce non solo alla riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento atmosferico, ma anche al miglioramento della qualità dell'aria nelle nostre città. Di fronte a questa opportunità non possiamo permetterci di ignorare il potenziale del telelavoro e dobbiamo lavorare insieme per creare le condizioni affinché questa modalità di lavoro diventi la norma e non l'eccezione. Ma come possiamo affrontare queste questioni in modo efficace e sostenibile? È fondamentale che il Governo collabori a stretto contatto con le controparti svizzere e con le parti sociali al fine di individuare soluzioni condivise per il telelavoro. Questo processo potrebbe includere la definizione di regole chiare e trasparenti in materia di orari di lavoro, responsabilità, diritti e obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché la garanzia di un adeguato sostegno tecnologico e infrastrutturale per agevolare il lavoro da casa. In conclusione, affrontare la questione del telelavoro per i lavoratori transfrontalieri tra Italia e Svizzera è di fondamentale importanza per garantire un futuro migliore e più equo per tutti i lavoratori coinvolti nonché per sostenere lo sviluppo socioeconomico nei territori di confine. Chiediamo al Governo di dare seguito a questo impegno e di trovare soluzioni adeguate al più presto. Nonostante l'attuale mancanza di una soluzione adeguata per il telelavoro, il provvedimento di cui discutiamo oggi rappresenta un traguardo importante per i lavoratori transfrontalieri e per i territori di confine tra Italia e Svizzera. Gentile Presidente, onorevoli colleghi, vorrei attirare un momento la vostra attenzione su un evento che per certi versi è storico di questa attività parlamentare. L'intervento che avete appena ascoltato non è mio. A dire il vero non è il prodotto nemmeno dell'intelligenza umana; è il prodotto di un algoritmo di intelligenza artificiale Chat GPT-4 ed è stato validato in collaborazione con una società di *engineering* che si occupa di intelligenza artificiale e di transizione digitale. Quanti di noi oggi sono in grado di distinguere un testo prodotto dall'intelligenza umana e un flusso di pensieri, che in ambito tecnico si chiama *chain of thought*, prodotto da un algoritmo di intelligenza artificiale? Questo intervento vuole essere una provocazione per aprire un dibattito pubblico serio in Italia, al di là delle mode del momento, per analizzare le implicazioni etiche, economiche e sociali dell'utilizzo degli algoritmi di intelligenza artificiale. La crescita dell'intelligenza artificiale è impressionante e può comportare grandi opportunità in settore economici strategici e nel progresso scientifico, ma può comportare anche rischi, in caso di utilizzo improprio e manipolativo nella diffusione di informazioni errate o nell'alterazione dei processi decisionali. Concludo l'intervento sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato e consapevole nei confronti dell'innovazione tecnologica che consideri sia l'opportunità che i rischi legati all'impiego dell'intelligenza artificiale affinché la tecnologia sia al servizio dell'uomo e del bene comune e non costituisca una minaccia per la nostra democrazia.

ratifica dell'accordo con la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri. Abbiamo esaminato un po' di tempo fa questo provvedimento proprio qui al Senato in prima lettura; un accordo che sostituisce quello del 1974, attribuendo i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. L'accordo definisce anche le cosiddette aree di frontiera, che per quanto concerne l'Italia sono le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, nonché la Provincia autonoma di Bolzano.

che hanno coinvolto dal 2019 le Province e hanno portato a superare le criticità dell'accordo che era stato siglato dal Governo Renzi nel 2015,

ad applicarsi il regime di tassazione esclusiva in Svizzera. A titolo di compensazione finanziaria, la Svizzera è tenuta a versare, fino alla fine del 2033, una somma a favore dei Comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Tra l'altro, nel provvedimento, oltre ai miglioramenti ottenuti grazie all'impegno della Regione Lombardia che ha superato determinate criticità, sono stati votati in prima lettura degli emendamenti della Lega a firma del presidente Garavaglia e sottoscritti anche da

dei lavoratori nei territori di confine: ciò per scongiurare la desertificazione produttiva, in queste aree di confine, dovuta alla maggiore competitività salariale dei territori oltre confine. Si tratta di risultati importanti, perché la possibilità di utilizzare questo fondo per gli assegni integrativi è un principio quella che può essere definita una zona economica speciale. Certamente bisogna fare molto per lavorare in questa direzione, ma è pur sempre un inizio. Ci tenevo a sottolineare questi emendamenti che sono stati approvati in prima lettura.

potesse siglare un accordo per il telelavoro; modifica che è stata inserita, motivo per cui oggi siamo qua a votare il testo definitivo. Ricordo inoltre, prima di concludere l'intervento, che abbiamo depositato sempre in quest'Aula alcuni ordini del giorno,

impegna il Governo a definire e affrontare meglio la tematica dello *smart working* e il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia che lavorano in Svizzera come frontalieri, ancorché ancorché in modalità di *smart working*. Poi, come dicevamo prima, sul tema della zona economica speciale, si chiede di rendere sempre più omogenea la capacità di competere da parte di questi territori, che sono le zone di confine rispetto ai territori svizzeri, attraverso l'istituzione di zone economiche speciali delle aree di confine, per quanto riguarda le Province di Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como e Sondrio, che sono anche oggetto di un disegno di legge che la Lega ha presentato sia nella legislatura

nella Regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, per favorire una presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto al di là dei confini istituzionali nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti. Infine, è stato chiesto un impegno al Governo affinché si attivi per far sì che venga ulteriormente implementata l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti. In quelle aree,

assolutamente favorevole al fatto che finalmente si arrivi alla definizione di questo Accordo, con le modifiche importanti che sono state introdotte sicuramente grazie all'intervento della Regione Lombardia e anche grazie a proposte emendative presentate dal

G12.2 a condizione che, al secondo impegno, siano anteposte le seguenti parole: «a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di». G12.3 è accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: dopo le parole «impegna il Governo» aggiungere le seguenti: «a valutare l'opportunità di introdurre rispettivamente»;

«impegna il Governo a tenere conto delle richieste di collaborazione che dovessero pervenire per ridare impulso alle attività della stessa istituzione, al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti». G12.5, il Governo lo accoglie a condizione che il dispositivo sia così riformulato: «impegna il Governo ad attivarsi affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera,

al primo impegno, espungere le parole «in modo da renderlo strutturale per il periodo successivo a giugno 2023»; al secondo impegno, sostituire le parole «ad attivarsi» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di attivarsi».

è evidente che non c'è la volontà di portare avanti la stabilizzazione dello *smart working*. Mi rivolgo anche al collega Romeo e al collega Garavaglia, che non vedo. che non vedo. Se il Governo annacqua gli ordini del giorno, anche quelli della Lega, che fa parte dello stesso Governo, mi sembra più una presa in giro che una reale volontà di risolvere il problema. Detto questo, accetto la riformulazione, ben consapevole del fatto che non affronterete il tema e che lo lascerete cadere fino al prossimo Governo.

Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra su un provvedimento che complessivamente risponde al bisogno di offrire una maggiore tutela ai lavoratori e alle lavoratrici, anche, ma non solo, in termini di fiscalità. Nello specifico, con questa ratifica andiamo a sostituire l'ormai vetusta normativa del 1974, che regolava solo il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavoravano in Svizzera. Ora, invece, andiamo a disciplinare anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia, nel segno quindi del principio di reciprocità. Si stabilisce un meccanismo di tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato fonte del reddito del lavoratore dipendente, in questo modo riconoscendo al lavoratore italiano un credito d'imposta per quanto versato in Svizzera. Questo ci sembra un passo nella direzione del pieno rispetto del principio di non discriminazione del lavoratore frontaliero nel trattamento fiscale. L'accordo è un atto dovuto per quei lavoratori e quelle lavoratrici che aspettavano da anni di godere di un regime diverso, in particolare sul terreno fiscale. Ribadisco poi all'Aula che stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici che hanno un salario discreto, quasi il doppio di quello dei lavoratori italiani. Sarebbe ora che questo Parlamento mettesse all'ordine del giorno, in cima alle proprie priorità, la situazione dei salari e delle condizioni di lavoro Vorrei innanzitutto che si prestasse attenzione e si svolgesse una discussione pacata - come l'ho sentita fare in questo caso e nelle scorse sedute sedute - ad esempio sul fatto che negli ultimi anni in Italia non basta lavorare per essere considerati fuori dalla povertà. Oggi anche un lavoratore rischia di essere povero. Sono tanti i lavoratori e le lavoratrici che non riescono a progettare un futuro. Vorrei, quindi, che la discussione sulle condizioni di lavoro questo Parlamento la svolgesse fino in fondo. Se, infatti, è stato facile metterci tutti d'accordo quando l'argomento all'ordine del giorno riguardava le condizioni di lavoratori con salari di una certa entità, molto più complessa è la discussione sulle condizioni di lavoro che riguardano milioni di persone che nel nostro Paese vivono la precarietà e sono sull'orlo della povertà. Sarebbe forse il momento di affrontare il grande tema del divario, che negli ultimi anni si sta acuendo, fra chi fra chi ha condizioni di privilegio, pochi, e chi scivola pericolosamente verso la povertà: tanti, purtroppo. Nell'annunciare il voto favorevole al provvedimento, chiedo quindi che venga data rappresentanza alla situazione in cui ci troviamo, una situazione in cui il lavoro è diventato sempre più povero e sempre più precario. Questo Parlamento dovrebbe avere la forza e l'onestà, anche intellettuale, di provare a dare una risposta che, in tutti questi anni, non è stata mai fornita. Deve diventare una priorità affrontare il fatto che, in Italia, i salari e gli stipendi dei lavoratori sono inadeguati. È necessario e non più rinviabile individuare un meccanismo che sia in grado di adeguare i salari

è un punto fermo che riusciamo a mettere dopo tanti, troppi anni, anche di controversie, tra l'Italia e la Svizzera. Esso è inoltre frutto di un lavoro fatto non solo da questo Governo, ma anche dal Governo precedente. Bisogna dare merito al lavoro che è stato fatto ed anche alla continuità che su questo punto si è voluto portare avanti in maniera opportuna. questioni importanti, che abbiamo già avuto modo di sottolineare. Penso ai profili sociali rispetto al tema dei lavoratori transfrontalieri; penso al coinvolgimento degli enti locali, in una meritoria opera di federalismo fiscale, che è stato fatto proprio affinché i Comuni delle aree al confine tra Italia e Svizzera possano offrire tutti quei servizi che consentano ai lavoratori transfrontalieri di svolgere al meglio le loro attività. Oggi poniamo un punto di termine di termine rispetto a un negoziato molto complesso, che ha affaticato il nostro Paese per tanti anni. Deve essere, però, anche un punto di partenza per tutte le questioni che ancora devono essere affrontate, alcune delle quali emerse nel dibattito di oggi e anche nel dibattito precedente che abbiamo avuto tra la Camera e il Senato. Io penso che tale ratifica ci debba avviare a una discussione bilaterale con la Svizzera, a favore e a tutela dei Comuni che si trovano ai confini e dei lavoratori transfrontalieri. Esprimiamo, dunque, un giudizio positivo sulla conclusione dell'accordo e voteremo favorevolmente.

la materia su cui oggi quest'Aula è chiamata a pronunciarsi necessitava da tempo di un intervento, che per la sua natura affronta questioni sostanziali, che interessano ed impattano sulla vita e la quotidianità di centinaia di migliaia di lavoratori frontalieri. È del tutto evidente di come precedenti accordi tra l'Italia e la Confederazione svizzera, risalenti alla metà degli anni Settanta, risentissero del trascorrere del tempo e del mutare delle condizioni e, pertanto, richiedessero una revisione che potesse regolare, per il presente e per il futuro, una materia tanto articolata quanto delicata con termini che potessero soddisfare i diversi *stakeholder* coinvolti ed interessati. Soprattutto, non possiamo non considerare che tale intervento si inserisce all'interno di uno sviluppo proficuo delle relazioni bilaterali tra i nostri Paesi, con una crescente collaborazione dei rapporti tra Berna e la stessa Unione europea che, come ci ricordano le parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della sua recente visita elvetica, vanno coltivati con ancora maggiore convinzione, poiché siamo *partner* necessari, affidabili, amici, interdipendenti, uniti da un destino comune dettato dall'appartenenza alla civiltà europea. Questi accordi sono quindi funzionali anche a rinnovare e a rinsaldare il nostro legame con la Confederazione; un rapporto strategico per il nostro Paese che, pertanto, va considerato anche oltre l'importante questione di confine, la cui implementazione risponde più che mai a ragioni di interesse nazionale. Non dimentichiamo infatti che l'Italia è uno dei principali *partner* commerciali della Svizzera, collocandosi tradizionalmente al secondo posto come Paese fornitore e al sesto posto tra i Paesi di destinazione dell'*export* della Confederazione, con un saldo commerciale in attivo e crescente. In particolare, la Svizzera rappresenta il quarto Paese al mondo per destinazione dell'*export* italiano, con una quota del 5,47 per cento del totale e figura al nono posto tra i Paesi di origine delle importazioni italiane. Il saldo commerciale a favore del nostro Paese è poi cresciuto in questi anni fino alla quota di 500 milioni di euro, raggiungendo i 16,1 miliardi. A questi dati economico-commerciali vanno associate alcune considerazioni di natura strettamente geopolitica e tutt'altro che secondarie. La Svizzera è membro di ventisette organizzazioni ONU, contribuisce al bilancio di altre dieci e partecipa ora, anche con unità dotata di proprio armamento, ad alcune forze internazionali di *peacekeeping* in aree per noi strategiche quali, ad esempio, il Kossovo, in cui in questi giorni e in queste ore si stanno consumando fatti inquietanti e drammatici. A tal

Comprendiamo tutti che, di fronte a questi numeri e a un *partner* così attivo in ambito multilaterale in teatri a noi prossimi e di interesse, le sollecitazioni che da tempo ci provenivano dalle autorità elvetiche affinché si aggiornassero gli accordi preesistenti che regolano i frontalieri non potevano essere ignorate e costituivano un terreno di azione e di confronto ineludibile anche al fine di tutelare i diritti dei cittadini italiani - di cui questi nuovi accordi tengono ampiamente conto - che giornalmente attraversano la frontiera per ragioni di lavoro. Non c'è dubbio

che, mi preme sottolineare, grazie al regime transitorio inserito nell'intesa siglata il 23 dicembre 2020, non subiranno alcun inasprimento degli oneri tributari dovuti, dopo che si è proceduto a modificare la prima versione della riforma stipulata con i negoziatori elvetici nel dicembre 2015 e ai quali si applicherà il regime di tassazione esclusiva in Svizzera. Tanto loro quanto i nuovi frontalieri che non risiedono nei Comuni di confine in futuro potranno dunque godere di uno sconto di 10.000 euro sul reddito imponibile in Italia, oltre ad ottenere la possibilità di dedurre dal reddito imponibile anche i contributi pagati sul salario per il prepensionamento e di portare a detrazione tutta una serie di spese (mutuo della casa, spese sanitarie, spese scolastiche, spese professionali di trasporto e via dicendo) che non vengono riconosciute nel sistema di tassazione alla fonte alla fonte oggi applicato dalle autorità fiscali elvetiche. Inoltre, si ipotizza per i frontalieri un'indennità speciale di disoccupazione, dimostrando così un'attenzione per tutti i lavoratori e in particolare per gli ultracinquantenni che, a a causa della crisi, si trovano senza occupazione e necessitano, quindi, di accedere agli ammortizzatori sociali previsti. Sono però due gli aspetti innovativi del nuovo Accordo che mi preme sottolineare. Il primo è l'inserimento della causa di reciprocità. Infatti, contrariamente alle disposizioni allo stato vigenti, è garantita la reciprocità di trattamento per i frontalieri italiani e svizzeri: le stesse regole vigenti per gli italiani che svolgono un'attività lavorativa in Svizzera varranno per i residenti elvetici che svolgono un'attività lavorativa in Italia. Si pone così fine a una disparità di trattamento che penalizzava in parte il nostro Paese, anche se non vi è alcun dubbio che il numero di transfrontalieri svizzeri è nettamente inferiore a quello dei transfrontalieri italiani; ciò anche a causa della scarsa appetibilità del nostro mercato del lavoro, su cui alcune forze politiche del nostro Parlamento farebbero bene a riflettere. Non si tratta, tuttavia, di un fenomeno trascurabile, poiché è crescente il numero di coloro che attraversano quotidianamente la frontiera italiana per ragioni di lavoro. Il secondo aspetto su cui mi preme soffermarmi è quello legato alle misure di sostegno finanziario per i Comuni di confine. Recepire le istanze di queste realtà territoriali è stato a mio avviso importante, non solo perché si salvaguardia per un decennio la compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ma perché anche in prospettiva si stabilisce di investire su tali realtà, non solo per favorire il loro sviluppo economico, ma anche per contrastare e ridurre quel fenomeno dello spopolamento, che purtroppo ben conosciamo, a cui sono soggette dette realtà. Onorevoli colleghi, l'Accordo che ci apprestiamo ad approvare, frutto di un lavoro che scavalla legislature ed Esecutivi - ne approfitto per ringraziare i colleghi di maggioranza e opposizione che vi hanno lavorato rappresenta quindi un testo ottimo per riformare le regole relative all'imposizione dei lavoratori frontalieri; per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune delle principali questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Lo spirito unitario che ha contraddistinto il suo *iter* parlamentare testimonia come le forze politiche siano ben consce della sua importanza. Lo siamo certamente noi di Forza Italia che, anche in questa sede, non possiamo che votare a favore della ratifica di questi accordi, ben sapendo che la riunione quinquennale di riesame bilaterale fra le due Nazioni, che potrà dettare modifiche all'Accordo e che prevede, insieme a un lungo e forse un po' farraginoso *iter*, anche l'intervento parlamentare, dovrà tener conto delle eventuali problematiche che dovessero emergere nel corso della sua esecuzione. Annuncio quindi, a nome del Gruppo cui appartengo, il voto favorevole a un Accordo che reputiamo equilibrato, nell'interezze di due Nazioni amiche.

che permetterà di superare il regime di doppia tassazione, archiviando così i vecchi accordi fiscali del 1974. Dopo anni di attesa, questa situazione è stata finalmente risolta e ne siamo soddisfatti. Peccato che ci sia invece una specifica situazione ancora irrisolta. Il MoVimento 5 Stelle, infatti, esprime forte rammarico e preoccupazione per la mancata soluzione definitiva del cruciale problema del lavoro da remoto dei nostri transfrontalieri; problema sul quale noi ci siamo impegnati per primi, seguiti da altre forze politiche di maggioranza e opposizione, ma non dal Governo, se non *in extremis* e in modo a dir poco limitato. Mi riferisco ovviamente al mancato rinnovo dell'Accordo sul telelavoro dei frontalieri, che era stato siglato dal secondo governo Conte nel giugno del 2020 in piena pandemia; un Accordo importante che il Governo Meloni, per dimenticanza o incuria, ha lasciato scadere a fine gennaio, creando gravissimi problemi di organizzazione familiare a circa 90.000 lavoratori italiani, per non parlare delle ripercussioni negative sul traffico stradale e inquinamento ambientale. Grazie al *pressing* politico del MoVimento 5 Stelle, iniziato nel corso della prima lettura qui in Senato, con la presentazione dell'ordine del giorno del collega Marton, il Governo si era impegnato ad avviare con urgenza i negoziati con il Governo della Confederazione svizzera. Ma il risultato è stato solo l'inserimento di una norma transitoria nel presente disegno di legge di ratifica, che prevede una proroga temporanea dell'Accordo sul lavoro da remoto con valore retroattivo per coprire il periodo successivo alla scadenza. Peccato che questa proroga scada solo tra un mese, il 30 giugno. Ciò significa che entro la fine di giugno è necessario trovare una nuova intesa per evitare che dal 1° luglio tutti i frontalieri siano costretti a tornare a tornare al loro posto di lavoro oltre confine per non incappare nei controlli del fisco italiano. Oggi torniamo quindi a chiedere con forza al Governo Meloni di impegnarsi per risolvere questo problema non con pezze temporanee o nuove proroghe, ma in maniera strutturale e stabile con il rinnovo dell'Accordo. La nostra richiesta è che il Governo concluda subito con la Svizzera un'intesa definitiva analoga a quella siglata mesi fa tra Svizzera e Francia, per cui il lavoro svolto a domicilio fino al 40 per cento del monte ore complessivo, ovvero due giorni a settimana, non metta in discussione lo *status* di lavoro frontaliero e conseguentemente non comporti penalizzazioni dal punto di vista fiscale e previdenziale. Oggi il MoVimento 5 Stelle voterà a favore di questa ratifica, con l'auspicio che il Governo Meloni e i ministri Tajani e Giorgetti non tradiscano le aspettative di decine di migliaia di famiglie e di lavoratori transfrontalieri che aspettano una soluzione definitiva e strutturale del problema del lavoro da remoto.

anche la soddisfazione per un percorso che si chiude dopo due anni e mezzo di lavoro; un lavoro importante portato con le realtà territoriali, con i sindaci dell'Associazione dei Comuni italiani di frontiera (ACIF), con il sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino, con le forze sociali e con i sindacati. Questo Accordo fiscale fra Italia e Svizzera l'abbiamo costruito con un approccio diverso rispetto al passato, quindi non *top-down*, calato dall'alto, ma *bottom-up*, e cioè coinvolgendo le realtà territoriali. a condurlo in porto con la piena condivisione dei soggetti territoriali è che per la prima volta questa si tratta non della semplice ratifica di un accordo stipulato tra due Paesi, ma del tentativo di costruire un approccio per ripensare le economie di confine. Le Province del Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio hanno nella parte di confine del loro territorio delle economie profondamente integrate,

E di questo siamo stati ringraziati, perché potevamo tenerli da questa parte del confine, in quella fase di emergenza che mordeva soprattutto nei territori della Lombardia colpiti prima di altri da quell'emergenza,

ristoranti ed esercizi commerciali, che si reggono proprio per il potere d'acquisto più alto degli svizzeri e che sono andati in crisi, in mancanza di clienti. a fronte di un sistema industriale e manifatturiero che subisce un costo del lavoro più alto rispetto a quello della Svizzera, con una tassazione molto più bassa. L'Accordo in esame prevede un bilanciamento e riconosce, per la prima volta,

della fascia compresa nei venti chilometri dal confine, che hanno costruito le proprie prospettive di vita e acceso mutui in base a un tipo di tassazione, quella svizzera, molto più bassa. Quindi la promessa «non un euro in più di tasse» è stata mantenuta. Allo stesso tempo, per i nuovi lavoratori frontalieri si prevede una tassazione più bassa, seppur più alta rispetto a quella dei vecchi frontalieri, perché innalziamo la franchigia.

risorse che sono state garantite anche per il futuro. In più - ed è la vera innovazione - costruiamo il primo esperimento di federalismo fiscale: l'extragettito delle tasse delle tasse che verrà pagato dai futuri lavoratori rimarrà sul territorio, su un fondo per lo sviluppo socio-economico e infrastrutturale del confine. È un riconoscimento della specificità di quell'area e di un'economia che si tiene in equilibrio in maniera molto

È il motivo per cui noi oggi torniamo a votare. Prevediamo una copertura retroattiva, da febbraio fino al 30 giugno di quest'anno, ma non basta. È un problema molto sentito nelle fasce di confine

rischiano di penalizzare dal punto di vista fiscale i lavoratori italiani che, rimanendo in Italia oltre un certo limite di ore lavorate, finiscono per pagare le tasse in Italia, con un aggravio molto forte rispetto al loro trattamento economico. l'emendamento che è stato approvato alla Camera e che oggi noi ci apprestiamo a ratificare in terza lettura. Occorre tuttavia che il Governo mantenga gli impegni, come noi abbiamo chiesto più volte. Siamo preoccupati che il ministro Giorgetti sia fortemente in ritardo nel ragionare con la controparte elvetica, perché dobbiamo dare un orizzonte futuro certo e di serenità a quelle famiglie che rischiano di avere un aggravio di molte centinaia di euro ogni mese sulla busta paga. Speriamo che

iniziato sotto la spinta del Partito Democratico due anni e mezzo fa e che oggi portiamo finalmente a compimento. colleghi, rappresentanti del Governo, nel ringraziare il collega Menia, che mi sta a fianco, esprimiamo particolare soddisfazione per ciò che oggi andiamo a votare. Votiamo un testo unificato, con la modifica, rispetto alla proposta precedentemente votata al Senato, dell'articolo 12, includendo - come ha detto il collega Alfieri - i lavoratori che operano in servizio presso il proprio domicilio, ovvero il cosiddetto lavoro agile e telelavoro: questo per noi è molto importante. I contenuti delle intese bilaterali sono destinati a riformulare a riformulare un'intesa attualmente in vigore, che risale al 1974, che a breve compirà più di cinquanta anni. Tali accordi sono frutto di un confronto decennale e di relazioni tra le parti interessate, vanno verso l'obiettivo di garantire il principio dell'equità fiscale, a noi particolarmente caro sempre, e non solo in questo caso. L'obiettivo elimina tutte le criticità sorte negli anni precedenti, evitando che i lavoratori che risiedono e lavorano in Paesi diversi siano soggetti a doppia imposizione fiscale. Ricordo che altre inequità similari sono presenti anche in altre realtà territoriali a noi vicine, quali la Francia e il Principato di Monaco, per citarne due, su cui auspichiamo azioni similari a quella che stiamo votando. Oltre a quanto detto, come è stato ribadito già precedentemente, il provvedimento in esame elimina le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. Mi preme però sottolineare che, proprio in un'ottica di semplificazione, che tutti continuiamo ad auspicare, e di trasparenza, viene introdotto il principio di cooperazione amministrativa, che attraverso la previsione di uno scambio di informazioni, quali dati identificativi dei lavoratori, dei dati sull'ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori, nonché di tutti i dati identificativi del lavoratore, consentirà allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, mediante un flusso elettronico verso la direttrice della digitalizzazione, di applicare la propria tassazione. mi piace sottolineare che assume particolare rilievo l'introduzione di una apposita disposizione volta a prevedere la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria, proprio in base a disposizioni contrattuali, che sono a carico dei lavoratori frontalieri. In base a tale previsione, i lavoratori potranno finalmente fruire della deducibilità dei contributi medesimi. Cruciale è l'esclusione dalla base imponibile Irpef degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa, che riguarderà però tutti i lavoratori frontalieri, poiché tali somme hanno natura non retributiva, bensì assistenziale. È per i motivi fin qui esposti che annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

L'ordine del giorno reca: «Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Cottarelli».

dopo aver ricevuto l'offerta, da parte dell'Università Cattolica di Milano, di andare a dirigere un programma di educazione nelle scienze economiche e sociali. Questo programma è rivolto agli studenti delle superiori di tutta Italia, copre tutto il territorio nazionale e consiste in visite da parte di personaggi che hanno una storia e una carriera a livelli elevatissimi per condividere con gli insegnanti e con gli studenti...

Questo programma consiste nella visita nelle scuole superiori di tutti Italia da parte di personaggi che hanno avuto una storia e una carriera professionale a livello altissimo, con lo scopo in parte di fornire informazioni nelle aree dell'economia e del diritto e nelle altre scienze sociali, ma sinceramente anche di ispirare insegnanti e studenti

ai cambiamenti climatici, di questioni relative al rapporto tra economia e diritto e alla Costituzione, nonché di una parte di comunicazione di queste politiche. È un programma che credo sia molto utile al Paese e ai nostri giovani. Purtroppo, è incompatibile con il lavoro di senatore, fondamentalmente per due motivi. Il primo è un motivo di percezione: il programma non può essere diretto da qualcuno che svolge un ruolo politico; il secondo motivo è pratico:

vado a dirigere questo programma, piuttosto che rimanere qui. Non credo di aver fatto male come senatore

di accettare le mie dimissioni già oggi, per un motivo ben preciso. Se si vuole far partire il programma su tutto il territorio nazionale nel prossimo anno scolastico, è necessario nel corso delle prossime

Non sempre sono d'accordo con lui, come egli peraltro sa, perché abbiamo avuto modo di discutere nel merito di alcune questioni nel corso dei mesi passati. Per storia, per biografia, forse anche per cultura politica,

penso che il contributo che il senatore Cottarelli ha portato al Senato della Repubblica in questi mesi sia stato davvero di grandissima rilevanza. Mi dispiace molto parlarne al passato, perché perché avrei sperato che questo contributo potesse durare fino al termine della legislatura; penso anche però che, dinanzi a una richiesta così precisa ed esplicita,

c'è stato un apprezzamento non retorico e non di circostanza, ma davvero molto grande e molto importante. Signora Presidente, anche il mio sarà un intervento molto breve. Desidero innanzitutto ringraziare Carlo Cottarelli per il contributo che ha dato all'interno della Commissione finanze del Senato in tutti gli interventi che ha svolto, perché è stato molto costruttivo, al di là dell'appartenenza specifica a un singolo partito. La seconda considerazione che voglio fare è che non è un buon segno per la politica se, dentro le istituzioni, non c'è spazio per il contributo di una persona come come Carlo Cottarelli. *(Applausi)*. Questo è un aspetto che pone un problema di qualità della politica e chi sta in quest'Aula ha il dovere di interrogarsi sul perché una persona di fatto lasci questo luogo. Ultima questione: noi, come Gruppo Per le Autonomie, asseconderemo la richiesta di Carlo Cottarelli, quindi voteremo a favore dell'accettazione delle sue dimissioni. Desideriamo comunque ringraziarlo per il contributo

Signora Presidente, la notizia delle dimissioni del senatore Cottarelli,

unito a una convinta speranza. Rammarico perché se ne va da quest'Aula una persona che ha dato un contributo molto importante alla vita pubblica italiana e al bene comune in Italia, ben prima di apparire in Senato. Per anni ha tenuto una posizione molto elevata e molto delicata. Per anni Carlo Cottarelli ha tenuto al Fondo monetario internazionale una posizione molto elevata e molto delicata, contribuendo al prestigio dell'Italia. Poi ha diretto, più di recente, un'operazione importante di *spending review*. Da un po' di tempo sentiamo meno questa espressione, ma non credo che il Paese senta meno tale esigenza.

non contestata da nessuno, è servita in un passaggio delicato della vita repubblicana. E poi, sia pure da poco, lo vediamo come senatore. La mia convinta speranza è che la voce del professor Cottarelli non si attenuerà. Cambierà sede, cambierà forma, ma non credo che il suo impatto sulla vita collettiva dell'Italia e sulla maturazione dell'opinione pubblica italiana diminuisca; anzi, penso che possa essere ancora superiore. Il senatore aver accettato questo programma di educazione alle scienze economiche e sociali. Sono sempre stato convinto che, più ancora che le immediate decisioni prese da Governo e Parlamento, nella vita di un Paese chi forma l'opinione pubblica abbia un ruolo ancora più importante nel facilitare la comprensione delle buone politiche da parte dei cittadini. Proprio questa mattina il governatore Visco, concludendo la sua ultima relazione come Governatore della Banca d'Italia, ha detto qualcosa che, ascoltandolo, pensavo si applichi perfettamente a questo passaggio nella vita del senatore Cottarelli. Diceva il governatore Visco problemi come la riduzione del debito pubblico o l'adozione di stili di vita coerenti con la difesa dell'ambiente richiedono che la società li comprenda e faccia propri, non perché "ce lo chiede l'Europa", ma perché ci schermano dai rischi e dischiudono opportunità. È a questo che va rivolta una nuova riflessione collettiva a tutti i livelli, per comprenderne l'importanza e decidere insieme come governarne gli effetti. Ebbene, le lezioni che da molti anni, con grande concretezza, il professor Cottarelli, poi senatore Cottarelli, ha dato alla comunità italiana sulle insidie del debito pubblico, nell'immediato, ma soprattutto per le generazioni future, secondo me, è e sarà negli anni futuri la componente molto importante di un'ulteriore maturazione della nostra comunità politica italiana dentro quella europea per rifuggire dall'irresponsabilità che si scarica poi sui nostri figli e nipoti. Quindi, Carlo, auguri per la tua ulteriore missione.

da questo incarico, che credo nell'ordinamento italiano sia l'unico dal quale non ci si può dimettere senza l'accordo di altre persone. Evidentemente voteremo a favore, però non posso negare che lo faremo con

di attività parlamentare, ha lasciato sicuramente il segno. Mi lasci dire, signor Presidente, che lo ha fatto, come ci ha anche raccontato oggi, senza cercare il conflitto, stando ai dati e ai fatti, quindi aiutando

di impegnarsi in politica e che davanti agli altri cittadini si impegnano a farlo per una legislatura: se una persona del suo calibro decide che non è quella la migliore delle modalità, forse c'è qualcosa che a noi che restiamo deve dare da pensare. Mi lasci dire un'ultimissima cosa. Il nostro rammarico deriva anche dal fatto che sappiamo di perdere un solido riformista, una persona che ha ispirato al riformismo e al pragmatismo tutta la sua attività, non soltanto politica,

trovare il momento per entrare in punta di piedi ed uscire, altrettanto in punta di piedi, da uno degli incarichi e una delle responsabilità più alti che possano essere attribuiti a una persona. È un momento nel quale il panorama politico ci dice che il disperato bisogno di riformismo, che credo abbia anche questo Paese, non riesce a trovare una sua espressione, non soltanto nelle istituzioni, ma anche nella politica, che si va sempre che si va sempre più polarizzando, a destra e a sinistra, su posizioni che si allontanano dal riformismo e tendono a diventare ideologiche e adottare spesso bandierine ideologiche. Il fatto che lei vada via e - me lo lasci dire - la sensazione che non vada via soltanto per questo altissimo incarico, che noi apprezziamo e per il quale le auguriamo davvero ogni bene e ogni successo, dà anche il sentore che ci sia un pezzo d'Italia che in questa

Quelle dimissioni a volte possono essere frutto di pressioni esterne e di condizionamenti che nulla hanno a che fare con la reale volontà di chi le presenta, quindi ritengo che sia un passaggio a fondamentale tutela del libero esercizio di chi rappresenta i cittadini in queste Aule. Il senatore Cottarelli ha ben spiegato le motivazioni, che in realtà non sono frutto di pressioni esterne, ma della voglia di dare un contributo al Paese in un'altra veste e in un'altra sede. Ovviamente gli auguriamo buon lavoro e voteremo a favore della sua proposta di dimissioni, ricordando il contributo di serietà, di professionalità e di grande competenza, anche se - come ha detto il senatore De Cristofaro - anch'io non sempre sono stato d'accordo con le sue ricette economiche, che però sono state certamente portate da con grande capacità e serietà, ha cercato di dare risposte al Paese.

svolto in questi mesi, continuo, quotidiano, puntuale, rigoroso e competente. Abbiamo apprezzato in questi mesi di lavoro comune quanto l'applicazione di quel rigore in diversi passaggi legislativi non faccia altro che migliorare il processo legislativo. Carlo Cottarelli lo ha fatto portando

dove ha diretto il Dipartimento affari fiscali. Non vorrei poi dimenticare, come ricordava il presidente Monti prima, i suoi contributi istituzionali, tra i quali anche quello di commissario straordinario alla revisione della spesa. Insomma, Carlo Cottarelli non è solo uno straordinario tecnico, ma ha dimostrato di essere un eccellente senatore della Repubblica; è un profondo liberaldemocratico e lo ringrazio per tutte le volte in cui ci siamo confrontati e abbiamo avvicinato alcune posizioni anche dentro la nostra comunità politica. Mi permetterà, signora Presidente, di ringraziare

in linea con il suo rigore e la sua storia, il senatore Cottarelli ha chiesto a tutti i Gruppi, ovviamente a partire da quello a cui appartiene, di confermare questa sua scelta. Mi permetterà anche, signora Presidente, di ringraziarlo ancora più caldamente, perché penso che questa scelta di Carlo Cottarelli, che ci impoverisce e ci toglie qualcosa (e lui lo sa, perché gliel'hanno detto tutti i componenti del Gruppo Partito Democratico), sia però un esempio per tutti coloro che invece, quando decidono di lasciare, dimenticano la comunità che ha consentito loro di entrare in quest'Aula e magari scelgono altre strade e

i migliori auguri di buon lavoro al senatore Cottarelli. Ovviamente, la Presidenza

dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 3.50,

10.0.1 e inammissibile l'emendamento 10.101. Dichiara altresì improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 9-*bis*.0.100, 9-*bis*.0.101

a nome del mio Gruppo, intervengo sugli emendamenti che si riferiscono a questo articolo. Lo faccio perché nel corso dell'esame in Commissione, con le nostre proposte e con vari emendamenti soppressivi e correttivi, abbiamo cercato di migliorare gli aspetti più critici del provvedimento. I nostri emendamenti tenevano conto delle molte audizioni svolte, ma purtroppo non sono stati accolti dalla maggioranza di Governo. Con l'emendamento 1.3, in particolare, abbiamo messo in evidenza come per dare correttezza e possibilità di attuazione al decreto fosse necessario prevedere adeguate risorse, che invece non ci sono, attraverso l'istituzione di un fondo per gli interventi urgenti per gli anni 2023, 2024 e 2025, partendo da un presupposto

che condiziona le nostre vite, e un dato oggettivo, di cui non possiamo che prendere atto. Ne è testimonianza la stessa cronologia del decreto in esame: quando è stato varato, infatti, la maggior parte dei bacini idrografici del Nord Italia, a partire da quello del Po, erano in piena siccità. Oggi, mentre siamo ancora in fase di conversione, il Parlamento è impegnato con un altro decreto ad affrontare le conseguenze dell'alluvione che ha devastato l'Emilia-Romagna e ha causato ingenti danni anche nelle Marche e in Toscana. È l'ultimo esempio che ci fa capire - con buona pace dei negazionisti in materia - che il cambiamento climatico è una realtà e che ricorda a tutti noi una volta di più quanto il nostro Paese sia fragile ed esposto a forti rischi idrogeologici, che continua a consumare una risorsa non rinnovabile e decisiva come il suolo. Di fronte a questo si dovrebbe comprendere da parte di tutti che l'unica strada percorribile è quella della transizione ecologica per approdare a un modello di sviluppo equo e sostenibile e che per impedire il ripetersi di simili tragedie il piano fondamentale su cui muoversi è quello della prevenzione. In tutto ciò ci ritroviamo a esaminare un provvedimento che, invece, non è all'altezza di questa situazione, figlio di un modo di legiferare improvvisato e tale da creare una serie di incoerenze, che credo vadano sottolineate. Quanto alla prima, in questi giorni abbiamo ascoltato il Presidente del Consiglio affermare più volte che la nomina del commissario per l'Emilia-Romagna non è una priorità. Dopodiché questo decreto si riduce di fatto alla nomina di un commissario straordinario nazionale *(Applausi)*, rispetto al quale peraltro si configura un ruolo non adeguato alla gestione di interventi che coinvolgono vaste aree sulle quali operano con compiti diversi enti territoriali diversi (ARERA, Autorità di bacino, consorzi di bonifica, altri commissari già incaricati di gestire le emergenze legate al controllo delle acque); per non parlare degli ingiustificati poteri attribuiti al commissario, visto che gli si consente di operare in deroga a ogni disposizione di legge, salvo quella penale. Si tratta di poteri sostitutivi che travolgono le competenze delle amministrazioni

andando a creare zone di incertezza e di conflitto istituzionale su una materia che, invece, necessiterebbe di un riordino, ma soprattutto di leale collaborazione. Intervenendo viene da commentare che a destra si vive - fatemelo dire - un'evidente contraddizione: da una parte, si predica autonomia; dall'altra, invece, con il dirigismo delle nomine e l'ipertrofia dei commissari, si pratica centralismo. Oltre a questo c'è un'oggettiva nebulosità su come si attiverà rispetto ai criteri con cui stabilire le priorità di intervento. Tutto, purtroppo, sembra essere lasciato al libero arbitrio, con un evidente quanto ingiustificato elemento di discrezionalità della cabina di regia del commissario: cosa preoccupante, se calata nella realtà. Penso alla deregolamentazione per la realizzazione delle vasche di raccolta di acqua piovana, senza precisare tra l'altro l'esclusione di opere di impermeabilizzazione permanente del suolo e l'utilizzo di cemento,

al PNRR qual è la posizione del Governo rispetto al tema della risorsa acqua, della salvaguardia del territorio e del controllo al dissesto, perché si tratta di interventi tutt'altro che marginali in relazione al ruolo e ai compiti del neocommissario. Tra le proposte del PD ce ne sono molte che potrebbero contribuire a migliorare il provvedimento e chiedo ancora ai colleghi di considerarle nell'ambito di questa fase di discussione, prima delle votazioni. Concludendo, mi soffermo sull'istituzione di un fondo straordinario per misure urgenti sulla rete fluviale. Si tratta di un fondo che ha come obiettivo la realizzazione di interventi per restituire spazio ai fiumi; per ampliare le casse di espansione; per ridurne la canalizzazione, ripristinando le connessioni tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo e modificando parte degli sbarramenti esistenti; per favorire interventi finalizzati alla ricarica degli acquiferi nel sottosuolo, nei periodi di *surplus* idrico. Insomma, l'accumularsi di grandi quantità di pioggia in pochissime ore, in territori fortemente antropizzati, impone interventi tempestivi e urgenti in questa direzione, per evitare di farci trovare impreparati a gestire al meglio situazioni di criticità. Insomma, ci saremmo attesi maggiori capacità di ascolto e di confronto da parte della maggioranza. Visti i pregressi, è vero che non si può restare troppo sorpresi se abbiamo trovato il solito atteggiamento di chiusura. Questa volta però il merito della questione - voglio dirlo, concludendo - avrebbe dovuto fare la differenza, permettendo per una volta di dimenticare le appartenenze politiche, mettendo al primo posto l'interesse generale, la cura del territorio e la vita delle persone. Molto probabilmente dobbiamo però tornare lì dove siamo partiti: la verità è che in ampi settori del Governo e della maggioranza il cambiamento climatico è sottovalutato e questa è la cosa più grave, perché significa non aver capito le criticità e i problemi del tempo in cui viviamo.

valutare l'opportunità di prevedere, per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, l'introduzione quale parametro di premialità di opere atte all'incremento della infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei».

Molte delle senatrici e molti dei senatori qui presenti sono stati amministratori locali e sanno quanto le amministrazioni comunali siano chiamate a svolgere la loro parte diligente e quanto siano coinvolte. In questo emendamento e nei

All'articolo 1 si prevede che venga redatto dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un decreto di ripartizione per i fondi che serviranno a emergenze su opere idriche. Mi chiedo come mai in questo decreto non venga interessato anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e questo si aggancia al discorso della spoliazione del Parlamento della sua funzione. Anche per l'emendamento 1.58 che andremo a votare tra poco la stessa richiesta riguarderà l'interessamento delle Commissioni competenti

se è possibile rivedere il parere, in quanto suppongo che non vi siano oneri finanziari scoperti che impediscano l'approvazione di questo emendamento. In tal modo si ripristinerebbe un dibattito parlamentare più intenso.

apportare un cambiamento al paradigma dell'utilizzo equo ed efficiente delle risorse. In questo caso specifico chiedevamo, nell'utilizzo degli invasi per uso di acqua potabile o per uso industriale,

Signor Presidente, di questo emendamento abbiamo discusso in Commissione e il Governo aveva detto che avrebbe fatto una riflessione. Insieme a vari Gruppi dell'opposizione, chiedevamo che la cabina di regia prendesse in considerazione anche il coinvolgimento delle università e dei centri di ricerca per utilizzare le migliori tecnologie e i migliori studi per il monitoraggio delle reti idriche. Possiamo davvero immaginare un decreto-legge sulla siccità in cui interveniamo senza sfruttare le conoscenze scientifiche, le università e i centri di ricerca del Paese, coinvolgendoli nel monitoraggio delle attuali reti e infrastrutture idriche?

chiedere supporto alle università italiane e ai centri di ricerca italiani per utilizzare la tecnologia per monitorare le reti idriche. *(Applausi)*. Chiedo che il Governo e i relatori possano spiegare a quest'Assemblea il motivo per cui si rifiuta di dare questa possibilità.

in dichiarazione di voto per spiegare anche il senso dell'emendamento. In questo decreto si parla di emergenza, necessità, velocizzazione, semplificazione e di tutto quello che serve per affrontare l'emergenza siccitosa in corso. serie di interventi e una serie di caratteristiche che vanno a contraddistinguere alcune figure individuate nel decreto. Quello che manca - a mio avviso - e per questo ho proposto l'emendamento, è l'individuazione di criteri specifici secondo cui andare a individuare la priorità degli interventi da porre in essere. L'emendamento in

avevamo previsto che, sentito anche il parere degli enti territoriali, il commissario potesse decidere di ridurre l'utilizzo dell'acqua potabile minerale per la vendita ad uso commerciale e quantomeno, che dall'approvazione del decreto, per le captazioni successive ci fosse una sospensione della concessione dello sfruttamento delle falde per questo tipo di acqua. Ecco perché chiediamo l'approvazione

ci tengo a intervenire su questo emendamento perché in Commissione abbiamo lavorato ascoltando molti soggetti,

Io penso che il Governo abbia sempre ragione, per definizione. In questo caso il Governo ci ha spiegato che anche se noi abbiamo recepito un suggerimento giusto da parte dell'ANCE, la stessa associazione non era informata del fatto che il nuovo codice degli appalti risolve questo problema.

senatore Sigismondi di Fratelli d'Italia e si è sbagliato. Abbiamo presentato tutti lo stesso emendamento, ma nessuno ha capito che questo problema era già risolto dal codice degli appalti. Considero giusto sottolineare che è increscioso che la più importante associazione nazionale che si occupa di appalti e di costruzioni non sia competente in questa materia. Il Governo fatto bene a bacchettarla bocciando questo emendamento.

Mi fa piacere che maggioranza, relatori e Governo abbiano apprezzato l'importanza della circolarità del ciclo dell'acqua, quindi delle acque sotterranee e del loro prelievo, ma soprattutto della loro ricarica.

si parla di investimenti, nel senso che per realizzare in modo oculato l'utilizzo e riciclo dell'acqua occorre investire in indagini e raccolta dati, in modo da poter avere il quadro della situazione e muoversi di conseguenza.

per far funzionare le pompe per prelevare l'acqua dei pozzi. È un'operazione energivora

di Treviso. Siamo tutti sensibili a ciò che mangiamo, ma credo che chi vuole sostenere soprattutto l'agricoltura del Nord sia interessato alla qualità delle acque. Tutto il decreto siccità si fonda su controlli *ex ante*. L'ordine del giorno G7.3 va semplicemente a potenziare i controlli *ex post* sulla qualità delle acque che andranno ad innaffiare

8a e 9a, che consente la sperimentazione in campo aperto di piante geneticamente migliorate grazie alle nuove biotecnologie agrarie. Credo sia un passo veramente importante per il Paese, ragion per cui vorrei sottolinearlo. È una notizia attesa dagli studiosi italiani e credo anche che sia un passaggio molto importante per quest'Assemblea che onora tutti voi; ma proprio per questo mi chiedo perché questo onore debba avere una data di scadenza. L'ultima riformulazione infatti aggiunge un limite temporale che trasforma questa norma importante in un'apertura mutilata, prevedendo che le disposizioni contenute nella norma valgano fino al 31 dicembre 2024. Ho chiesto i motivi dell'inserimento di questa data, ma non ho avuto precise spiegazioni. Credo che sia giusto pensare a una norma ponte, nell'attesa della disciplina europea, ma proprio per ma proprio per questo non serve mettere una data finale; quando interverrà l'Europa, la norma italiana semplicemente verrà meno. Il problema del non rimuovere la data è che, appunto, questa diventa una norma mutilata, un'apertura mutilata sotto diversi profili. sotto il profilo scientifico, perché chiunque faccia ricerca sa che un anno e mezzo di tempo è troppo breve per sviluppare pienamente un progetto, soprattutto quando si tratta di studiare le rese di colture in campo aperto. Chiunque fa ricerca sa bene che i bandi pubblici chiedono almeno due o tre anni di sperimentazione, quindi il ricercatore sarebbe mutilato, anche

Aggiungo che l'apertura è mutilata anche considerando i benefici sociali ed economici che si vogliono ottenere con la norma, in quanto gli effetti dei cambiamenti climatici che si vogliono che si vogliono contrastare con la norma (pensiamo alla siccità) non cesseranno di certo tra un anno e mezzo; quindi non è davvero congruo inserire un termine temporale. A me sembra mutilata anche dal punto di vista legislativo, perché già oggi sappiamo che si dovrà comunque intervenire nuovamente dal punto di vista normativo, visto che il tempo non è sufficiente. È mutilata anche dal punto di vista culturale, perché si dà un messaggio pessimo. Il messaggio è che basta comprimere i tempi amministrativi entro i quali si chiede alla ricerca e agli studiosi una soluzione, per avere le soluzioni; non funziona così. Per questo ho presentato un emendamento che lascia intatto l'impianto dell'articolo ed elimina solamente il termine del 31 dicembre 2024,

di una disciplina organica in materia da parte dell'Unione europea. Mi sembra che eliminare quella data sia il modo migliore per onorare il vostro lavoro, quest'Aula e per riconoscere la capacità dei nostri ricercatori.

molto delicato in questo Paese, ossia l'agricoltura geneticamente modificata. Come ben sa la senatrice Cattaneo, in questo Paese è vietato l'OGM. Io ho fatto un intervento, in Commissione, dicendo che, personalmente,

questa, una ipocrisia tipicamente italiana. È anche vero, però, che in questo Paese ci si divide tra contrari e favorevoli su tante forse anche senza approfondire. Ricordo, ad esempio, la battaglia contro l'agricoltura biologica e biodinamica; anche in quel caso la scienza non è venuta molto incontro a chi, invece, voleva un'agricoltura più

con piante diverse, in modo tale che quella più fragile raccoglie la forza di quella più forte. Quindi, si tratta di qualcosa di completamente diverso dall'OGM, ma è comunque una sperimentazione in ambito agricolo.

campagna di *fake news* contro la possibilità che, anche nel nostro Paese, si arrivasse all'OGM. Questo anno e mezzo, che alla senatrice Cattaneo sembra un tempo molto breve, in realtà serve a fare una campagna informativa per minare *a priori* le *fake news* che, che, ahimè, determinerebbero ancora una volta un nulla di fatto, come purtroppo è avvenuto nella passata legislatura. Lo splendido lavoro svolto dal presidente Gallinella non un deputato o un senatore di Italia Viva, ma del MoVimento 5 Stelle, non è purtroppo riuscito ad approdare a un contributo fattivo, cioè ad una legge (perché noi siamo qui per fare le leggi, non per fare dibattiti), proprio per la preventiva bocciatura pubblica

aprirebbe un dibattito eccessivamente violento contro una pratica che invece deve finalmente approdare a un risultato definitivo. In questo caso ci aiutano i progetti di legge depositati e che chiedo al presidente Luca De Carlo di calendarizzare calendarizzare al più presto possibile, in modo che in questo anno e mezzo arrivino a conclusione sia alla Camera che al Senato. come Alleanza Verdi e Sinistra, riteniamo inopportuno, inappropriato e fuori luogo che nel decreto-legge sulla scarsità idrica si parli di autorizzazioni per le emissioni deliberate nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico, che dovrebbe fornire indicazioni agli agricoltori. Paradossalmente, in tutto il decreto-legge sulla crisi idrica non si è ritenuto di entrare nel dettaglio di tecniche volte a ridurre lo spreco di consumo d'acqua nel settore industriale, agricolo e domestico. Eppure, stranamente e improvvisamente, emendamento decontestualizzato da ogni logica intrinseca a questo decreto. Prima di proporre tali emendamenti bisognerebbe discuterne ampiamente in Commissione sulla base di una seria ed approfondita base documentale, anche perché trattano temi delicati su prodotti che vengono equiparati agli OGM e assimilabili a varietà derivate da mutazioni naturali o selezioni tradizionali. Bisogna discuterne chiedendo delle audizioni in merito che possano estendersi a tutti i corpi intermedi e alle associazioni coinvolte. Come ho già detto ieri sera in discussione generale, è importante non essere frettolosi finendo per fare male, ma sentire tutte le parti coinvolte e partire subito bene. ragioni, dichiaro il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra su questo emendamento, evidenziando anche con dispiacere che il mio voto di astensione rispetto all'emendamento sull'*editing* genomico, votato ieri in Commissione, non è stato rilevato.

sicuramente cambiare idea fa parte delle sue prerogative e quindi accettiamo la sua astensione, anche tardiva. Dico una cosa molto semplice: le tecniche di evoluzione assistita non sono OGM, e questa è una premessa che va fatta in maniera chiara. Sono tecniche fondamentali per lo sviluppo dell'agricoltura, ma rappresentano un tema molto delicato si presta a parecchie strumentalizzazioni fuori da quest'Aula. All'interno di quest'Aula, e nella fattispecie in Commissione, siamo riusciti - grazie al lavoro di tutti, mio, del senatore Paroli che ha presentato un emendamento simile al mio, del senatore Bergesio che pur non avendo presentato un emendamento è sempre stato anche in Commissione un grande fautore di queste tecniche, del senatore Centinaio - a far percepire, anche a quelle parti politiche che oggi non sono la maggioranza e che quindi avrebbero potuto astenersi o votare in modo contrario rispetto a questi temi, l'importanza delle tecniche di evoluzione assistita. Lo abbiamo fatto spiegando che questo emendamento ha un termine temporale, perché nelle more di questo anno e mezzo

quanto tale tematica sia approfondita dal Parlamento, perché ne conosce le fragilità e le criticità. Lo abbiamo fatto tutti assieme, perché siamo convinti del ruolo centrale del Parlamento (quindi delle Commissioni) e ieri sono stato particolarmente orgoglioso che questo che questo testo fosse votato da tutti. In questo anno e mezzo noi ci dedicheremo, proprio in Commissione, a licenziare un provvedimento senza un termine temporale che sia frutto del lavoro parlamentare e che consenta al nostro Paese di porsi in maniera avanguardista anche rispetto alla nuova agricoltura, sapendo benissimo che su questo è importantissimo, come diceva prima la senatrice Fregolent, non solo agire, ma anche saper comunicare, per evitare di fare di tutta l'erba un fascio e per evitare che le tecniche d'evoluzione assistita con gli OGM. Anche l'Europa ha capito che non è questo il caso; io, infatti, mi confronto parecchio con l'onorevole De Castro e abbiamo la stessa visione su questo tema. Sappiamo che l'Europa è indietro rispetto a questa tematica, perché quando nascono le TEA ha già legiferato per gli OGM,

dimostreremo al Paese quanto sono importanti le TEA e lo faremo con un approccio assolutamente partecipativo, che consenta a tutti di potersi esprimere, ma anche di rendersi conto di quali differenze ci sono tra le *fake news* e la realtà. *(Applausi)*.

9-*bis*.100 ci sia un invito a fare veloci per la sperimentazione, per l'approfondimento, per l'attività di comunicazione necessaria su un tema essenziale e su cui si possono ingenerare anche dei fraintendimenti come quello attuale. Pertanto noi raccoglieremo anche in Commissione

togliere un limite temporale per questa attività e per questo elemento necessario a chiarire tutti gli aspetti e a comunicarli nei modi opportuni. Per questo noi ci asterremo sull'emendamento.

confermano la grande potenzialità di questa tecnica. Nell'ordine del giorno in esame ho inserito la possibilità di garantire le coltivazioni nei campi attigui, con una forma di assicurazione in caso

sicuro della bontà di queste forme sperimentali e quindi esonerandolo da ogni eventuale rischio.

non ha, come per il resto su altre misure, una visione unitaria né organica. Con questo emendamento ci siamo permessi, come Gruppo, di proporre un Piano nazionale per definire una strategia unica che possa permettere di affrontare in maniera adeguata, pesata e ponderata tutte le azioni future,

proposta di modifica integrale all'articolo 10 dà anche la possibilità al Governo di rivedere questa posizione: abbiamo veramente intenzione di governare questo processo, che è legato ai cambiamenti climatici? Lo vogliamo fare in maniera oculata, facendo i giusti passi? Perché non partire da un Piano nazionale, dando la possibilità a organismi già costituiti

adeguare gli impianti esistenti anche dal punto di vista degli impatti energetici. Ci accingiamo a votare, in ambito di Unione europea, un aggiornamento di direttive, tra cui quella legata agli impianti di potabilizzazione o comunque agli impianti di acque reflue in generale. L'Unione europea ci dice in maniera chiara che dobbiamo adeguare gli impianti di depurazione esistenti perché sono eccessivamente energivori, perciò entro il 2040 anche gli impianti esistenti devono

questo approccio, che siano impianti neutrali dal punto di vista delle emissioni carboniche e siano indipendenti dal punto di vista energetico. Porto a conoscenza, Presidente, per il suo tramite anche al Governo,

derivanti dalla dissalazione. Per perorare la causa proposta giustamente anche dal collega Lorefice, nell'emendamento 10.15 chiediamo di ridurre l'area entro la quale è possibile che la variazione della salinità della salinità sia superiore al 5 per cento, così come definito dal decreto in oggetto. Chiediamo di ridurre

o comunque dove non vi siano aree sensibili o dove vi sia la presenza di maree capaci di mescolare la quantità salina immessa in mare e ciò semplicemente per tutelare l'ambiente, anche perché non sappiamo che impatto avremo con le nuove disposizioni. Chiedo al Governo di riflettere su queste proposte, che certamente non spostano denari, ma vanno a creare un ambiente più tranquillo. Ovvero, nel momento in cui andiamo a creare questa serie di dissalatori, vogliamo prevedere un piano per omogeneizzare la presenza dei dissalatori nei nostri territori, chiedendovi almeno un occhio di riguardo su quelle che saranno le condizioni degli scarichi che avete individuato per le salamoie.

immettere acqua buona, pagata a caro prezzo, in reti bucate, con perdite di oltre il 50 per cento. Secondo me è un controsenso e pertanto l'abrogazione di quei commi della legge salva mare sono o

che io penso potrebbe essere congrua al nostro bisogno come Paese è la realizzazione dei dissalatori. Ci sono già delle ipotesi in alcune città; per esempio, la città di Genova si è già candidata ad ospitare una soluzione di questo tipo. Esistono degli approfondimenti rispetto alla quantità di risorse che sono utili a questo tipo di infrastruttura e anche di impianti che potrebbero soddisfare un'articolazione del problema del Paese sul tema della siccità; più o meno sette-otto impianti. Penso che noi dovremmo prenderci un impegno serio - mi rivolgo al Governo - sia nella direzione della progettualità legata ai dissalatori che della quantificazione del numero di impianti necessari. Continuiamo a parlare di infrastrutture e a dire che in questo Paese il tema del cambiamento climatico - lo dico anche con riferimento a quello che è accaduto in Emilia-Romagna sia solo parzialmente risolvibile con un intervento di modificazione, per esempio, dei temi del consumo del suolo. Certo che ci vuole anche una strategia strategia correttiva su questo piano, ma poi ci sono delle situazioni che non saremo mai in grado di risolvere se non ci doteremo di impianti, infrastrutture ed interventi in grado di risolvere strutturalmente il problema. Lo stesso vale per la siccità. È inutile girare intorno ai temi: abbiamo bisogno di grandi infrastrutture che mettano a disposizione quelle realtà che si sono già in qualche modo candidate e rese disponibili per il Paese. In queste ore c'è una discussione infinita sul PNRR, con il tentativo di tirare da una parte e dall'altra, affermando che un Governo è stato più o meno capace di un altro. di mettere in campo idee nuove e progetti diversi; facciamo qualcosa perché in questo Paese non si pianga sempre il giorno dopo in cui la siccità prevale e il giorno dopo in cui le alluvioni arrivano e spazzano via interi territori. A me piacerebbe chiedervi

con un indirizzo serio e credibile perché questo Paese la smetta di piangere il giorno dopo in cui gli eventi sono arrivati e i problemi si sono palesati.

Signora Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, mi sia concessa un'amara riflessione: sembra quasi che il destino si faccia beffa dei lavori parlamentari.

intervento? Chiedo contestualmente ai colleghi che vogliono abbandonare l'Aula di farlo molto celermente e anche silenziosamente.

Oggi in quest'Aula parliamo di siccità e crisi idrica, mentre in questi stessi giorni si continua a spalare fango, a mettere in sicurezza persone e strade, si continua a piangere le vittime dell'immane tragedia che ha colpito al cuore l'Emilia-Romagna e tutti i suoi cittadini, a cui rinnovo tutta la mia solidarietà e vicinanza. Il paradosso della siccità: mai così tanta acqua in trentasei ore in quella regione. Si potrebbe proprio sintetizzare con questa affermazione la calamità che si è abbattuta sull'Emilia-Romagna, una calamità in grado di riversare su quei territori oltre 350 milioni di metri cubi d'acqua per 800 chilometri quadrati di territorio, che hanno coinvolto 100 comuni, ben 23 fiumi e 13 corsi d'acqua. Con questo paradosso nel cuore, bisogna però dire che la siccità non è più un'emergenza, ma ormai è diventata un problema strutturale e ciclico, un problema che però, per la prima volta nella storia del Paese, questo Governo di centro-destra ha deciso di affrontare concretamente e con un decreto *ad Un problema di natura emergenziale se si guarda all'anno 2023, ma che va letto in chiave strutturale se si considera che negli ultimi vent'anni il 2023 è il quinto anno nel quale si verifica un evento siccitoso e le alluvioni si moltiplicano da anni. Lo dico chiaramente, signor Presidente, senza timore di smentita: nessun Governo fino a questo momento aveva scelto di affrontare la crisi idrica in modo davvero strutturale, checché ne dica il PD. L'impatto del cambiamento climatico sul settore primario è devastante, con danni quantificabili in diversi miliardi Le norme che il Governo Meloni con lungimiranza ha inserito nel decreto siccità all'esame di quest'assise vanno quindi nella giusta direzione. Si tratta di norme per la prevenzione e il contrasto della siccità e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni delle risorse idriche. Tutto ciò non rende comunque l'idea di quello che avrebbe dovuto essere fatto in passato e che, invece, con ogni evidenza, non è stato fatto; quello che doveva essere affrontato da chi fa della transizione ecologica il proprio *mantra* e l'unico obiettivo dell'azione elettorale propagandistica, da chi vede nel PNRR la soluzione a tutti i disastri e attribuisce ad altri i ritardi della sua attuazione. Presidente, il cambiamento climatico è forse la causa primaria di certe calamità, ma le ragioni profonde di quello che è accaduto in Emilia Romagna sono forse da ricercare altrove. Le rilevazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) parlano chiaro. Ciò significa che si sarebbe potuto e dovuto intervenire prima, senza smantellare ciò che di buono avevano fatto alcuni Governi. Parlo, ad esempio, senza remore di «Italia sicura» del Governo Renzi. E invece non si è intervenuti e oggi ci troviamo di fronte a quello che viene definito il paradosso dell'acqua: siccità, eventi climatici calamitosi, innalzamento dei con tutto quello che a questi fenomeni consegue in termini di dissesto idrogeologico e conseguente pericolo per le popolazioni e per l'ambiente. Non dobbiamo, anzi, non possiamo lanciare un messaggio infarcito dei soliti slogan propagandistici; così come non possiamo negare che il sistema climatico sta ciclicamente cambiando e che questi cambiamenti abbiano naturali Per quanto riguarda l'acqua, ad esempio, non bisogna considerare solo i prolungati periodi di siccità; al contrario, come, purtroppo, si è plasticamente verificato nelle zone emiliano-romagnole, spesso anche le piogge, che a lungo mancano, si riversano a volumi torrenziali in periodi molto concentrati, sicché ai danni da siccità vanno ad aggiungersi quelli ingentissimi da inondazione. È quindi del tutto evidente che da quelle acque il territorio nazionale va protetto per evitare dissesti. Al tempo stesso, però, le acque vanno recuperate perché non vadano disperse. Presidente, è di palmare evidenza la fragilità del nostro bellissimo territorio italiano. Guardandolo dall'alto, possiamo renderci conto di come è caratterizzato: per un terzo da campi coltivati, per un altro terzo da boschi, laghi e fiumi, e per il rimanente terzo da insediamenti urbani e industriali. Due terzi di questo Paese rappresentano la bellezza che lo caratterizza, ed è proprio di questi due terzi che ci dobbiamo occupare. C'è bisogno di manutenzione, di infrastrutture e di raccolta delle acque per consentirne l'utilizzo anche in tempi diversi. C'è bisogno di efficientamento dell'esistente e di introduzione di nuovi strumenti. Anche in Anche in questo campo, come in molti altri, occorre un impianto normativo più snello e meno farraginoso, che non disperda in mille rivoli e pastoie burocratiche le direttrici e le azioni di intervento. C'è bisogno di sostenere le categorie produttive, sulle quali i problemi climatici impattano di più, e che colpiscono indistintamente il nostro Paese, da Nord a Sud, *in primis* il comparto agricolo. l'acqua, da annoso problema, si può trasformare in opportunità. Dobbiamo infatti sfruttare al meglio i giorni di pioggia che - voglio ricordarlo - sono circa 93 all'anno, che, attraverso i vasi e i canali di raccolta delle acque piovane, possono diventare fonti preziose di risparmio idrico civile. Onorevoli colleghi, è evidente che non è più pensabile l'idea di affrontare l'emergenza senza programmazione. Ciò che si rende assolutamente necessario è promuovere politiche della prevenzione attraverso la definizione di una strategia idrica nazionale, che abbia un approccio circolare con interventi di breve, medio e lungo periodo. Lo sviluppo dell'economia circolare è essenziale se si immagina, ad esempio, che nel nostro Paese non esiste un piano nazionale per il riuso delle acque da depurazione, di cui già semplicemente il 30 per cento potrebbe essere impiegato soltanto nel settore agricolo, mentre oggi viene disperso nei fiumi, nei laghi o nei mari. Una fotografia davvero impietosa in Italia: gli investimenti nel settore idrico sino ad oggi sono pari a circa 49 euro *pro capite*, a fronte di 100 euro impegnati in Europa. Investire sulle reti idriche è un obiettivo primario se si ha contezza che l'Italia è sostanzialmente ferma alle stesse capacità di invaso di mezzo secolo fa, ma con necessità e consumi aumentati enormemente. A chi ancora oggi continua a farsi portavoce portavoce di un ambientalismo meramente di facciata, ricorrendo ai soliti *slogan* recuperati da vecchi copioni elettorali, e che comunque - ricordiamolo - ha governato in passato, andrebbe fatto notare che l'Italia paga regolarmente pesanti sanzioni all'Unione europea per effetto delle diverse infrazioni in materia di infrastrutture idriche. Non dobbiamo poi dimenticare che il bacino idrico del nostro Paese ha una sua prospettiva storica. Non dobbiamo certo dimenticare che siamo il Paese che ha inventato gli acquedotti e i sistemi irrigui. Come non possiamo dimenticare che siamo i grandi realizzatori delle bonifiche; vantiamo imprese nazionali specializzate nel disinterramento di dighe e invasi, che, però - ahimè - come spesso accade, lavorano, con grande stima, all'estero. Se è vero che le misure adottate al Governo con il decreto-legge oggi in conversione porteranno benefici già nel breve periodo, è altrettanto vero che riteniamo essere necessari anche ulteriori interventi, come ad esempio la realizzazione di una rete di piccoli invasi con basso impatto paesaggistico, diffusi sul territorio, e ancora di una rete di micro e medi impianti per la raccolta delle acque piovane e fluviali, utilizzando senza sprechi e in modo attento e mirato i fondi del PNRR. Altrettanto necessario sarà agire sugli accordi di Basilea, tenendo conto delle particolarità dell'agricoltura, per prevedere interventi sulle procedure di istruttoria e deroghe apposite per il merito creditizio delle imprese agricole, rafforzando e facilitando il rapporto tra gli istituti di credito e le stesse imprese agricole. Sul piano ambientale dobbiamo evitare ostacoli al corso naturale dei fiumi, favorire il rimboschimento e garantire un uso razionale delle risorse d'acqua sotterranee. Dobbiamo anche ottenere dall'Europa deroghe all'uso non produttivo dei terreni e alla rotazione annuale obbligatoria dei seminativi. Il problema non sono certamente né i "nasoni" di Roma, né le "vedovelle" di Milano, posto che siamo i più alti consumatori *pro capite* di acqua in Europa, con oltre 220.000 litri al giorno per abitante, pagando il prezzo dell'acqua più basso d'Europa, un prezzo che certamente non disincentiva la cultura dello spreco. Presidente, vale la pena rimarcarlo ancora una volta: questo decreto-legge ci ricorda le tante azioni che possono e devono essere messe in campo e traccia una rotta che insegue non le sirene dell'ideologia, ma i dettami del pragmatismo nella gestione delle infrastrutture, nella prevenzione dei dissesti, nella salvaguardia dell'ambiente, nella tutela delle persone e nell'accompagnamento di filiere vitali, come quella agricola, verso un futuro che sta cambiando intorno a noi e che dobbiamo saper affrontare, preservando le nostre peculiarità e le nostre tradizioni e sfruttando le potenzialità dell'innovazione. Bisogna pensare a come utilizzare le nuove tecnologie per poter riutilizzare l'acqua anche per produrre energia, a maggior ragione pulita, come quella idroelettrica. A questo proposito, Presidente, non posso non rimarcare con forza gli emendamenti che avevo presentato a questo provvedimento, che renderebbero al Governo Meloni il riconoscimento

e di supportarne la piena e consapevole attuazione sull'intero territorio nazionale. Concludo, Presidente. C'è un modo di concepire l'ambiente come un vero e proprio atto di civiltà, un patrimonio da lasciare intatto ai propri figli e ai propri nipoti. Niente danze della pioggia, ma sblocco immediato delle opere e pianificazione, misure serie e concrete da attuare per dare soluzione ai problemi come mai nessuno è stato capace di fare. Con le azioni contenute in questo decreto-legge il Governo Meloni sarà capace di passare dalla teoria alla pratica, dalle parole ai fatti. Per questi motivi argomentati, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-MAIE ha dato e continuerà a dare il proprio contributo e oggi voterà

che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo prevedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lombardia a seguito delle dimissioni del senatore Carlo Cottarelli, ha riscontrato, nella seduta odierna, che la candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Cristina Tajani. Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatrice Cristina Tajani.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi assistiamo alla discussione e alla votazione dell'ennesimo decreto-legge che interviene in un'ottica emergenziale su un problema strutturale e cronico nel nostro Paese, che è collegato alla crisi climatica e i cui eventi estremi stanno colpendo ripetutamente l'Italia. Le immagini sono sotto gli occhi di tutti; occhi che purtroppo il Governo non è ancora disposto ad aprire per intervenire alla radice del problema. Nei sette mesi e mezzo del suo lavoro, il Governo non ha posto le basi concrete per affrontare in modo strutturale l'emergenza climatica che sta investendo l'Italia e che si manifesta con ondate di siccità e inondazioni di drammatica portata. È un triste dato di fatto che il Governo non abbia messo in cima alla propria agenda politica il contrasto agli effetti del cambiamento climatico. Non ce n'è, infatti, traccia nei provvedimenti che sono stati affrontati e approvati in questi sette mesi e mezzo. Non ce n'è traccia nemmeno nel decreto oggi in discussione, recante disposizioni urgenti per il contrasto alla scarsità idrica. In Commissione abbiamo ascoltato decine di esperti e professionisti, proposti trasversalmente da tutti i Gruppi parlamentari. All'unisono hanno attestato dati oggettivi sui fenomeni climatici e sui cambiamenti che stanno interessando l'Italia e presentato valide proposte rispetto al loro efficace contrasto. Avrei, quindi, piacere di sapere su che fonti si basa l'intervento del collega della Lega, il senatore Cantalamessa, quando ieri sera, con le sue parole, ha messo in dubbio la conoscenza scientifica, etichettandola come ideologica, favorendo così, di fatto, la diffidenza nei confronti della scienza e mettendo in dubbio l'evidenza scientifica. Milioni di dati che vengono incrociati, osservazioni satellitari, strumenti ad altissima precisione, database che vengono utilizzati per misurare e monitorare il clima e i cambiamenti climatici: e qui in Aula si mette in dubbio la veridicità di questi dati e la professionalità di chi li va a studiare. su quali fonti? Io trovo molto preoccupante cercare di scardinare il valore della scienza, cosa che non fa altro che fomentare quella sfiducia e quella diffidenza già diffuse nella società in diversi settori. È grave fare leva sulla paura rispetto all'incerto, allo sconosciuto, invece di rassicurare sul fatto che la scienza sia arrivata ormai a livelli di conoscenza e tecnologia che le permettono di indicare le soluzioni alle sfide che dobbiamo affrontare e non negarle. Ecco probabilmente il motivo per cui il Governo non ha ancora messo in campo una valida strategia per affrontare il contrasto al dissesto idrogeologico e agli effetti del cambiamento climatico. Manca la consapevolezza su come affrontare questa tematica complessa ed è evidente la mancanza di volontà di agire immediatamente per il bene del Paese Paese e delle comunità. Ritengo frustrante dover ripetere ancora una volta che l'aumento della temperatura media globale di 1,1 gradi rispetto all'era preindustriale è correlato agli eventi che stanno colpendo anche il nostro Paese, che sono sotto gli occhi di tutti. Ma veramente dobbiamo continuare ad ascoltare, anche in quest'Aula, colleghi che ci propinano ragionamenti negazionisti, come abbiamo sentito anche ieri dai banchi della maggioranza? Sembra che non bastino neanche le immagini tangibili dei danni che stanno causando gli eventi climatici estremi, che costano purtroppo la vita a numerose persone. Pensiamo solo agli ultimi eventi in Emilia-Romagna, a Ischia e nelle Marche. Ciò è inaccettabile nel 2023. Ieri sera mi sono arrivati anche i video del violento temporale e della devastante gradinata a Torbole sul lago di Garda, con le strade invase da acqua e ghiaccio. Chi vive in quei territori come me sa di cosa sto parlando. Sa che il mondo fuori è cambiato. Sono tutte immagini che fanno capire la dimensione dei danni ambientali e sociali, che stanno mettendo in ginocchio l'economia di interi territori. A quando un vero cambio di rotta da parte del Governo? Le soluzioni proposte dal decreto in discussione non tengono conto di tutte queste considerazioni e purtroppo fungono di nuovo da cerotto rispetto a un'emorragia in atto. Non sono soluzioni risolutive. Rispetto a questo decreto sulla crisi idrica oggi in discussione noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo detto sì all'inserimento di un comitato scientifico in pianta stabile nella cabina di regia. Il Regolamento europeo del 2021 (normativa europea sul clima) ci impone di istituire un comitato consultivo scientifico sui cambiamenti climatici. Il Governo ha detto no. Lo ha escluso, evidenziando un *modus operandi* carente di visione lungimirante e di conoscenza scientifica, che sono basilari per una efficace gestione della siccità e, più in generale, della crisi climatica in atto. Abbiamo detto sì all'inserimento in cabina di regia, in modalità definitiva e continuativa, degli enti territoriali preposti alla gestione della risorsa idrica, delle autorità e degli istituti scientifici centrali e locali, che nelle audizioni hanno chiesto esplicitamente un coinvolgimento attivo e costante. Il Governo ha detto no. Questo causerà seri corti circuiti a livello locale e forti rallentamenti nell'applicazione della norma. Abbiamo detto sì all'approccio partecipativo e inclusivo degli enti territoriali, le vere sentinelle del territorio italiano. Il Governo ha detto no: un vero controsenso se si pensa alle mire autonomistiche di parte di questo Governo. Abbiamo detto sì alle sacrosante richieste dei territori che chiedono il potenziamento, la formazione e la riqualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche locali, per dare manforte nel sostenere, monitorare e avviare un'azione sostenibile, inclusiva, condivisiva e partecipativa. Il Governo ha detto no. In questo modo si rendono complesse la prevenzione, la manutenzione e la gestione di soluzioni operative efficaci per affrontare la siccità. Abbiamo detto sì a collegare le misure della cabina di regia con il rispetto dei tempi e le modalità di attuazione dei progetti del PNRR, ma il Governo neanche l'ha considerato. È un fatto preoccupante alla luce anche dei dati divulgati in questi giorni dalla Corte dei conti sull'utilizzo inesistente delle risorse finanziarie finanziarie destinate alla transizione ecologica (sono stati utilizzati infatti solo 2,2 milioni); Corte dei conti alla quale il Governo adesso vuole porre il bavaglio, fatto altrettanto preoccupante. Abbiamo detto sì all'efficiente gestione ordinaria della risorsa idrica e soprattutto alla corretta applicazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e della direttiva alluvioni 2007/60/CE. Il Governo ha detto no. È grave non prevedere la manutenzione delle reti di distribuzione delle acque a qualsiasi uso, non adoperarsi anche per la loro digitalizzazione e ridurre ad esempio le perdite di acqua potabile, che in Italia arrivano fino al 45 Abbiamo detto sì alla promozione di metodi e di tecniche di risparmio idrico nei settori industriale, terziario, agricolo e anche domestico. Il Governo ha detto no. Ricordo che siamo il Paese che in Europa spreca più acqua e che investe meno sull'infrastruttura idrica. Abbiamo detto sì al mantenimento della procedura di valutazione di impatto ambientale. Il Governo ha detto no. È grave l'idea di eliminare la valutazione di impatto ambientale; in questo modo si segue una logica contorta, ma che noi tutti ben conosciamo. La convinzione diffusa è che, per fare presto, si devono bypassare procedure importanti per un territorio fragile come l'Italia, creando una giungla di eccezioni su eccezioni. Si pensa di semplificare e velocizzare, mentre invece si complica tutto ancora di più, compromettendo la realizzazione e la buona riuscita delle opere, allungandone paradossalmente i tempi. diciamo sì a fare le cose bene da subito per mettere in sicurezza il territorio. Il Governo dice invece no e anche in questo decreto-legge continua nella logica dell'eccezionalità che ha bloccato l'Italia; continua ad applicare deroghe su deroghe che impattano sui procedimenti e creano le basi per le scappatoie che, di fatto, danneggiano quel territorio e quell'ambiente che si deve poi andare a mettere in sicurezza quando il danno ormai è fatto. Noi diciamo convintamente sì ad affrontare e risolvere le cause di questi eventi climatici estremi con nuovi modelli gestionali e soluzioni innovative, in modo sistemico, strutturale e anche culturale. Governo dice convintamente no, limitandosi a rincorrerne i sintomi con risposte estemporanee ed emergenziali. Nel decreto-legge in esame non si interviene in un'ottica di prevenzione e si evita la manutenzione e l'ammodernamento di infrastrutture idriche già esistenti. Si preferisce inserire nuove opere, con il rischio reale di utilizzare progetti da anni dimenticati nel cassetto e con il mondo fuori che è cambiato. Abbiamo aspettato veramente tanto per questo decreto e siamo alle porte dell'estate, in un'Italia preda di alluvioni e siccità. Il risultato è deludente e dispiace prenderne atto. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra rinnoviamo l'appello al Governo a dire sì a una seria politica di contrasto alla crisi climatica. Rimettete in sicurezza l'Italia e la vita delle persone che vi abitano.

Signor Presidente, per l'Italia il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre, con un calo delle precipitazioni del 45 per cento. Coldiretti ha stimato un danno per il settore agricolo di 6 miliardi di euro. Non va meglio l'anno 2023: si prospettano danni al settore di 8 miliardi e un aumento del prezzo di alcuni prodotti agricoli fra il 10 e il 30 per cento. Ma c'è di più: i terreni disseccati e le colline spogliate dagli alberi per via degli incendi estivi non riescono ad assorbire le acque degli eventi atmosferici estremi, invadendo i campi e i centri urbani - è quello che abbiamo drammaticamente visto in Emilia-Romagna e nelle Marche a settembre - oppure provocano frane come quella che ha colpito la Val di Fassa in Trentino il 5 agosto dello scorso anno. Davanti a un quadro così drammatico è apprezzabile la volontà del Governo di introdurre norme per contrastare le disparità di risorse idriche e semplificare la costruzione delle opere per la messa in sicurezza del territorio. Tuttavia questi obiettivi, per essere raggiunti, devono vedere il massimo coinvolgimento degli enti regionali e locali, perché sono quelli che meglio hanno il polso della situazione e quindi la priorità da attribuire ai vari interventi. Sul punto riteniamo che il continuo ricorso alle figure dei commissari straordinari, a cui vengono attribuiti ampi ed eccezionali poteri, a prescindere dagli ordinari meccanismi (sicuramente migliorabili) e dai principi di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, desta non poche preoccupazioni per noi rappresentanti delle autonomie territoriali. In questo senso sarebbe stato opportuno che nella cabina di regia entrassero anche i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome direttamente interessate, anche in ragione delle competenze legislative e amministrative loro proprie in materia. Inoltre, anche in termini più generali, una eccessiva centralizzazione può deresponsabilizzare gli enti territoriali, inibendo lo sviluppo di un *know how* per fronteggiare la crisi ambientale. Semmai, per noi la questione è opposta: come sviluppare in ogni articolazione istituzionale la sensibilità e gli strumenti validi per la gestione delle acque, si tratti di siccità o di alluvioni. Da questo punto di vista è importante che nei lavori di Commissione il Governo abbia accolto alcuni emendamenti volti a limitare l'approccio centralista. Mi riferisco in particolare alle diverse modifiche volte a salvaguardare le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano sull'utilizzazione delle acque degli acquedotti e delle opere idrauliche.

Il Gruppo per le Autonomie esprimerà quindi un voto complessivamente positivo, anche se a nostro avviso permangono alcune criticità che auspichiamo possano essere superate in futuro. Il nostro voto è principalmente anche un invito a proseguire con sempre maggiore decisione sulla strada della prevenzione, della tutela del territorio e di politiche in grado di rispondere all'emergenza siccità. Signor Presidente, con il decreto-legge siccità si cerca di risolvere un'emergenza che ha attanagliato il nostro Paese per diciotto mesi consecutivi. Oggi che abbiamo un'alluvione alle porte forse ci siamo dimenticati di cosa ha l'estate più siccitosa accompagnata da un autunno siccitoso, accompagnato da un inverno siccitoso e di nuovo da una primavera siccitosa. Devo dire che le

sciistiche delle montagne, in un inverno in cui ha nevicato veramente molto poco. Il provvedimento in esame non risolve l'emergenza siccità, forse perché è arrivato così tardi; probabilmente non si volute mettere delle risorse vere per ristorare tutti i danni economici che le categorie hanno subito; esso fa un passo in avanti verso l'istituzione di un commissario e di una cabina di regia. Mi fa piacere che la collega Biancofiore abbia voluto sottolineare come ItaliaSicura sia stata l'ultima unità di missione, l'ultima cabina di regia dove

fossero del clan evviva Renzi. Ciò significa che effettivamente, con i dati alla mano, l'unità di missione ItaliaSicura è stata l'ultima

dà degli spunti positivi: cercare, in questo periodo, di abbreviare le tempistiche per alcune infrastrutture, in particolare sui dissalatori, sull'utilizzo e sul riuso delle acque grigie, sulla possibilità di fare bacini idrografici.

invece, si utilizzano le acque grigie, ovviamente depurate e opportunamente controllate. Perché in Italia, invece, questo non avviene? Ricordo, banalmente, che nei nostri water c'è l'acqua potabile e non l'acqua grigia, come avviene per esempio in Germania, in Francia e nel Nord Europa. Perché l'acqua costa poco. È impopolare dirlo. Bisogna invece dire che l'acqua costa, che bisogna farla costare ancora di meno, che ci deve essere il livello minimo gratuito per tutti, come se fossimo in Africa o nei Paesi più lontani dove l'acqua effettivamente è un'emergenza. Mi auguro che questa crisi idrica abbia

sono di nuovo foriere di una stagione nella quale si pensava che l'acqua fosse eterna. Il PNRR stanzia delle risorse, anche se non tantissime rispetto ad altre categorie, come la transizione energetica - se pensiamo a quanto utilizzato per per l'energia e quanto utilizzato per l'acqua, c'è una sproporzione - ma queste possono essere l'inizio di un'inversione di tendenza, per cui l'acqua viene utilizzata in maniera diversa per l'agricoltura,

all'altezza. Abbiamo votato contro tutti i provvedimenti in cui si negava un vero bacino, dove si prevedevano bacini senza l'uso di cemento, e non perché amiamo il cemento, ma perché i piccoli laghetti probabilmente servono per farci pascolare le papere, ma non per risolvere il dramma della siccità.

che nel prossimo decreto ci siano risorse certe per un settore come quello legato all'agricoltura, anche se ce ne sono tantissimi e non c'è soltanto il mondo agricolo in attesa di risposte concrete. Penso che nel prossimo decreto, che purtroppo vedrà un segno completamente opposto, visto che si parlerà di alluvioni - sembra folle, ma è così - ci sarà anche un'attenzione a creare un fondo legato alla crisi climatica. Per anni ci si è sforzati a dire che coloro che lo denunciavano erano fautori di

questa missione, partendo proprio dai cambiamenti climatici presenti in tutto il mondo e che devono avere come conseguenza delle scelte radicali,

all'aiuto delle opposizioni, riescano a vedere un cambio di rotta: meno emergenza e più programmazione. Lo chiediamo infine per l'ultima volta: rimettete la struttura di missione ItaliaSicura, *(Applausi)*, esattamente come avete approvato con ordine del giorno, perché quella cabina di regia è stata dichiarata da tutti l'unico e l'ultimo momento in cui il Paese ha speso sulle risorse idriche. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge di cui stiamo trattando, cosiddetto siccità, prevede misure per aumentare l'efficienza e la capacità dei sistemi idrici di resistere ai cambiamenti climatici che generano fenomeni meteorologici opposti. Ed è questo, colleghi, il tema che si vuole affrontare con questo provvedimento: l'effetto sul territorio dei cambiamenti climatici che, purtroppo, purtroppo, generano lunghi periodi di siccità e periodi di forti precipitazioni piovose che in poche ore concentrano la pioggia di mesi. L'alluvione di alcune province dell'Emilia-Romagna ha reso evidente nella sua tragicità il tema della gestione dell'acqua. Si tratta sicuramente di un intervento normativo urgente e, anche se lo si non è orientato solo alla risoluzione di questa vicenda - appunto quella della siccità - che causa enormi problemi alla produzione agricola, vista la carenza di bacini idrici e invasi. Ma è anche uno strumento adatto ad affrontare fenomeni meteorologici avversi cui abbiamo assistito più volte negli ultimi anni; non è una cosa nuova. Il largo apporto di memorie e contributi iscritti arrivato alle Commissioni ambiente e industria del Senato, che hanno esaminato il decreto, ha mostrato quanto vaste e parcellizzate siano le competenze in materia di gestione e raccolta dell'acqua in Italia. Sappiamo bene, colleghi, che è in atto un riordino in tutte le Province e in tutti i territori, ma è evidente che bisogna fare più in fretta: bisogna fare in modo che tutto ciò che si sta facendo si faccia più velocemente. Quindi ora il decreto tende a porre ordine alla materia, innanzitutto istituendo una cabina di regia per la crisi idrica presso la Presidenza del Consiglio. questo è un modo per cui il coordinamento di tutte le attività dei tanti soggetti pubblici, ma anche privati, coinvolti nella realizzazione e gestione delle infrastrutture idriche possano avere un'unica regia, un coordinamento, un punto di riferimento certo ed efficace.

Questi soldi andranno spesi in modo puntuale, posto che due miliardi di euro sono destinati a nuove infrastrutture idriche; 900 milioni di euro sono indirizzati alla riparazione, digitalizzazione e monitoraggio integrato delle reti, per diminuire le perdite d'acqua. sono destinati alla risoluzione di uno dei principali problemi della gestione dell'acqua nel nostro Paese, visto che le perdite superano in media il 42 per cento del totale immesso. perdite non nuove anche in altri Paesi: in Italia non siamo gli unici ad avere questa problematica, ma certamente non ci piace avere dei *record* su temi Avrebbe poco senso continuare a pompare acqua in acquedotti colabrodo: questo lo sappiamo bene, è già stato detto e bisogna fare in modo di evitarlo. Ulteriori 800 milioni di euro sono destinati al potenziamento e all'ammodernamento del sistema irriguo, a servizio dell'agricoltura. Altri 600 milioni di euro sono finalizzati agli investimenti per gli impianti di depurazione di acque reflue, che possono essere riutilizzate sia in agricoltura che dall'industria manifatturiera. Quindi, visto che le risorse economiche ci sono, bisogna risolvere gli ulteriori problemi, che sono quelli della selezione dei progetti più appropriati e fare in modo che dai progetti, opportunamente scelti per la loro realizzabilità, si passi ai cantieri e alle opere realizzate. Talvolta capita che acquedotti e depuratori vengano trattati anche dai territori che li devono ospitare, quasi come fossero centrali nucleari. Non si capisce il beneficio che questi impianti possono portare e se ne vede solo il fatto che possono disturbare, ma non si sa bene cosa. Di conseguenza, anche la semplificazione delle procedure di affidamento delle gare appare opportuna, perché c'è la necessità di fare bene, ma - come ho già detto - c'è anche Ci sono poi le norme per favorire la manutenzione degli invasi, posto che si estende la disciplina semplificata alla gestione dei sedimenti che derivano dalle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento. Questo è un tema su cui bisognava intervenire, perché finora questi materiali sono stati trattati come rifiuti - purtroppo non è l'unico caso - mentre al contrario sono e sono sempre stati risorse per l'edilizia, che possono e debbono essere riutilizzate al meglio. Vorrei ricordare che molte delle soluzioni proposte da questo decreto erano state proposte già nella scorsa legislatura da Forza Italia, che aveva presentato un proprio piano per la gestione dell'acqua. In molti casi ci si è trovati, fino ad oggi, di fronte a carenze di progettazione o di realizzazione degli interventi. Il decreto contiene molte proposte per velocizzare le procedure, superare il dissenso e mettere in atto i poteri sostitutivi in caso di inerzia e ritardo - su questo bisogna essere molto più drastici - così come prevede la nomina di un commissario nazionale straordinario, che ha e avrà il compito di monitorare lo stato degli interventi e adottare gli atti che ritenga necessari all'esecuzione dei progetti. La necessità è quella di utilizzare al meglio, cioè in modo efficace ed efficiente, i volumi di acqua per i vari scopi, ovvero l'agricoltura, l'industria, l'uso civile e l'idroelettrico. Sempre sul versante delle semplificazioni, ci sono misure per facilitare la realizzazione di vasche di raccolta di acque per uso agricolo, che potranno essere compiute in edilizia libera; così come sono semplificate le disposizioni per la gestione delle acque reflue e dei fanghi di depurazione. Sull'esempio di Israele, che da decenni utilizza l'acqua di mare per la propria agricoltura, sono adottate anche norme per la più celere realizzazione degli impianti di desalinizzazione, cosa della quale non dobbiamo avere timore. Insomma, il decreto contiene una serie di norme, di cui ci ha riferito in maniera puntuale il nostro relatore, il senatore Rosso, che ringrazio, che si propongono di utilizzare al meglio le risorse in campo. Lo scopo è completare, sì, i progetti già in fase di attuazione, ma anche realizzare i nuovi e facilitare la realizzazione da parte dei privati di tutte quelle infrastrutture che possono ottimizzare l'utilizzo dell'acqua. Apprezziamo inoltre che siano stati approvati alcuni nostri emendamenti e quindi ringrazio i relatori e il Governo. Un emendamento dispone che gli interventi e le attività relative alla realizzazione delle infrastrutture idriche siano considerati di pubblica utilità, come deve essere. L'altro prevede che per garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche possano svolgere in prossimità delle stesse attività di pulizia del materiale flottante con oneri anche di smaltimento a carico del gestore o del concessionario. Altra modifica accolta reca misure per favorire l'*editing* genomico (di cui si è parlato prima all'interno di emendamenti che abbiamo affrontato) in ambito agrario, prevedendo lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolari intensità, e biotici di particolari intensità, di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici. Non dobbiamo avere timore della ricerca, dobbiamo affrontarla in modo responsabile, ma anche puntuale.

siamo nuovamente in Aula a votare un decreto-legge del Governo. A votare, lo sottolineo, e non a discutere, parlare e dibattere. A questo Governo infatti il dibattito parlamentare non piace, evidentemente lo trova superfluo, come abbiamo detto e ripetuto tante volte in questa Aula e fuori; questa occasione ne porta un'ulteriore testimonianza. Nei lavori di Commissione i Gruppi di opposizione hanno avuto contezza delle inammissibilità sui propri emendamenti troppo tardi per poter riformulare proposte che potessero superare tali inammissibilità. Ciò ha di fatto precluso alle opposizioni di partecipare in maniera costruttiva ad una parte del dibattito parlamentare nel procedimento legislativo. La cosa che però colpisce ancora di più è il vuoto normativo e di contenuti nel quale fluttuano gli interventi ritenuti necessari ed urgenti da parte di questo Governo. Lo abbiamo visto

In sintesi possiamo dire che questo Governo si scaglia contro i percettori del reddito di cittadinanza, mentre garantisce ed assicura potere ai suoi attraverso il reddito di militanza. *(Applausi)*. proprio così perché l'unico obiettivo e risultato concreto che questo Governo sta portando a casa è la sua battaglia ai canoni d'arredamento: lotta al divano e passione sfrenata per la poltrona! *(Applausi)*. Di nuovo complimenti! Di nuovo!

Io non vi nascondo che inizialmente la cosa faceva ben sperare, sembrava davvero esserci stata una presa di posizione sull'importanza dei cambiamenti climatici, soprattutto da parte di quanti di quanti negazionisti siedono tra le fila della maggioranza. La verità però è che la *governance* ambientale di questo Paese sta dimostrando di essere inadeguata ad affrontare le problematiche in atto. Il decreto-legge annunciato è arrivato dopo oltre un mese e, una volta letto il testo, scusatemi, ma purtroppo ogni speranza si è rovinosamente sciolta come neve al sole, per restare in tema. Cosa fate infatti con questo decreto-legge? Voi identificate un'emergenza e mettete a gestirla un commissario un altro, l'ennesimo - e gli date sei mesi di tempo per realizzare un cronoprogramma di interventi su opere che gli verranno indicate dalla cabina di regia. Bene, ma stiamo parlando di opere che sono già previste e finanziate a legislazione corrente, senza aggiungere un euro per l'emergenza e soprattutto senza garantirne gli effetti positivi per il breve periodo.

un 2022 che si è contraddistinto come un anno nero per il discorso idrico. È stato uno dei più caldi e secchi e ha registrato il 50 per cento in meno di neve caduta e quasi il 50 per cento in più di fabbisogno energetico. Siamo alle solite: quest'Aula, dopo aver licenziato un provvedimento sul ponte che non parla di ponte, ora si trova a licenziare un provvedimento sulla siccità che non provvede all'emergenza della siccità in corso. A poco servono, cari colleghi, le vostre rassicurazioni, scritte nere su bianco, della proroga del commissario. A poco serve, soprattutto dopo che nella relazione tecnica che accompagna il decreto-legge avete sbagliato addirittura a conteggiare il compenso da corrispondere a questo povero commissario: la solita confusione che solo voi sapete fare quando si parla di necessità e di urgenze, perché anche qui, quando si parla di necessità e urgenza, lo stato confusionale è evidente e atavico. Purtroppo, ormai non ci stupisce più, lo capite? È questo il problema, ormai non ci stupite più. Soprattutto, Presidente, c'era bisogno di tante risorse in questo provvedimento, ma voi non le avete previste. Le uniche risorse che avete previsto sono quelle per il commissario e per la sua struttura, formata da dodici unità e cinque consulenti, i quali non avranno il problema del compenso per fortuna, ma avranno un altro problema, problema, ovvero non sapranno dove andare a lavorare. Non avete previsto una postazione lavorativa per loro: non una scrivania, non un ufficio. Ma come pensate di dare un incarico così importante a dei tecnici, senza pensare che queste persone dovranno recarsi in un ufficio per andare a lavorare, senza fornire loro la dotazione necessaria per poter lavorare per voi? Come si poteva intuire ed era prevedibile, anche questa volta i tecnici del servizio bilancio hanno sollevato delle criticità su questo decreto, ma a voi poco importa. Il Ministro, erede del Brunelleschi, ha detto che non si può perdere tempo in costi e benefici di opere e provvedimenti. D'altra parte, quando i conti non tornano - e a voi capita spesso - ve la prendete con la Corte, che è chiamata a vigilare sugli stessi.

possa avvenire solo su fondo naturale, senza l'uso di materiale edilizio, sia in virtù di una generale salvaguardia dell'ambiente, ma anche per l'alimentazione della ricarica in falda, ma a voi tutte queste cose non interessano. Siete andati dritti con la liberalizzazione, senza tra l'altro nemmeno giustificare il mancato gettito che ne deriverà per le casse dello Stato. È tutto riportato nelle note allegate al testo. All'articolo 10, invece, avete trovato la soluzione alla crisi idrica con i dissalatori. Lo fate ovviamente stravolgendo il lavoro che il MoVimento 5 Stelle ha fatto per difendere gli ecosistemi marini e costieri da questi impianti - ricordiamolo - energivori ed impattanti. Lo fate con modifiche puntuali legge "salva mare", eliminando quello che invece dovrebbe essere un passaggio propedeutico all'attivazione di qualsiasi dissalatore, ovvero la manutenzione sulla rete idrica esistente. Che senso ha velocizzare la proliferazione di questi impianti, addirittura escludendoli dalla VIA, cosa per noi imprescindibile, se poi una volta messi se poi una volta messi in funzione questi dissalatori non faranno altro che pompare nuova acqua in una rete che già oggi perde oltre il 40 per cento della materia immessa? Fatemi dire che tutto ciò ha davvero poco senso, soprattutto al netto di ulteriori osservazioni, come ad esempio quella che riguarda gli scarichi delle salamoie, che derivano dal processo di desalinizzazione. Avete definito che la variazione massima di salinità del corpo recipiente non può superare il 5 per cento della media nel raggio di 50 metri della zona dello scarico. Io voglio ricordare a quest'Aula - e prima di tutto a me stessa - che l'elevata salinità di un'area produce la riduzione del livello di ossigeno nell'acqua. La riduzione del livello dell'ossigeno nell'acqua impatta notevolmente sugli *habitat* marini, generando effetti osservabili lungo tutta la catena alimentare. Anche su questo ci auguriamo che siano state fatte delle giuste valutazioni e che non ci sia stata la solita confusione, perché se così non dovesse essere, ci ritroveremo a gestire problematiche aggiuntive. Vi stiamo avvisando. Vi abbiamo chiesto di modificare il testo della norma che avete scritto con accorgimenti di assoluto buonsenso, come quello di ridurre il raggio entro cui questa variazione di salinità viene consentita. Ancora, vi abbiamo chiesto di collocare gli scarichi a 200 metri dalla costa, lontano da aree sensibili, dove comunque viene garantito il ricambio delle acque che è in grado di disperdere i prodotti reflui derivanti dagli impianti di desalinizzazione. Ma a voi non è interessato né dibattere, né approfondire questi argomenti. Questo modo di agire, anziché risolvere i problemi, rischia di crearne altri. Signor Presidente, concludo. Questo provvedimento certifica ancora una volta l'inazione del Governo Meloni e la totale mancanza di visione programmatica e politica di questo Esecutivo. Nel caso specifico, la cosa non ci sorprende, come dicevo prima, visto che in tanti al Governo e in maggioranza non vedono nei cambiamenti climatici un'emergenza da gestire e da affrontare nell'immediato. Per questi motivi, Presidente, dichiaro il voto contrario del MoVimento 5 Stelle a questo provvedimento e al vuoto che lo riempie.

ci ricordano quanto distruttivi possano essere gli effetti del cambiamento climatico sul territorio, sulle abitazioni, sulle imprese, sulle infrastrutture. In brevissimo tempo, un territorio pesantemente colpito da due anni di siccità, con le portate dei fiumi ai minimi di sempre e l'avanzamento del fronte di intrusione salina per chilometri all'interno della fascia costiera, ha dimostrato con drammatica evidenza la sua fragilità dal punto di vista idrogeologico. Vasti allagamenti in pianura e rovinosi eventi franosi nella media collina hanno sconvolto la vita di migliaia di persone, causando la perdita di 15 vite umane e la morte di migliaia di animali, devastato case e imprese, distrutto raccolti agricoli e allevamenti, messo in serio pericolo l'inestimabile patrimonio culturale e artistico di cui è ricco il territorio alluvioniato. Credo che un doveroso ringraziamento vada rivolto alle forze della Protezione civile, ai numerosissimi volontari, prontamente intervenuti a salvare vite e cose *(Applausi)*, agli angeli del fango, subito in attività a supporto di quanti sono stati colpiti, a spalare melma e rifiuti da case e strade; ai consorzi di bonifica per il loro indispensabile contributo a limitare l'entità dell'impatto alluvionale, azionando pompe idrauliche e sistemi di convogliamento accelerato delle acque alluvionali attraverso i canali irrigui in mare, salvando così una parte importante del territorio. Oggi abbiamo tutti la consapevolezza dolorosa che molto è andato perduto per sempre, ma sappiamo anche che possiamo e dobbiamo contrastare i drammatici effetti del cambiamento climatico sul nostro territorio, con azioni decise e coraggiose, a tutela della risorsa idrica, per prevenire fenomeni estremi quali alluvioni e siccità, i cui effetti sono già evidenti e continueranno - per diversi anni a venire ad avere impatti sul contesto socio-economico e ambientale del Paese. I danni all'ambiente, all'economia, in particolare all'occupazione agricola, sono di milioni di euro, andandosi a sommare a quelli della siccità, che fino a metà maggio aveva compromesso la semina e il ciclo colturale di alcune produzioni. Il Governo, con il provvedimento che oggi andiamo ad approvare, fornisce risposte concrete a una situazione emergenziale, mai affrontata prima con forza e decisione come oggi, attivando tutti gli strumenti possibili per contrastare gli effetti della crisi idrica sul territorio, sull'ambiente, sulle comunità civili e sui sistemi produttivi, *in primis* sull'agricoltura. Abbiamo lavorato in modo responsabile, puntando sulla creazione di un sistema di *governance* efficiente, con il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti, tra cui le Regioni e le Province autonome, le Autorità di bacino la cabina di regia, che avrà l'importante compito di fare una ricognizione e una rimodulazione delle risorse attualmente disponibili e non ancora impegnate, andando a individuare in particolare le opere e gli interventi di urgente realizzazione ad opera poi di un commissario *ad acta*, ai fini dell'adeguamento della rete infrastrutturale idrica. Questo permetterà non di impiegare risorse aggiuntive, bensì di ottimizzare quanto già nelle disponibilità delle amministrazioni competenti. abbiamo detto più volte, tra le sue misure più caratterizzanti questo provvedimento ha il compito di aumentare i volumi idrici invasati, di semplificare le procedure per la realizzazione di infrastrutture idriche, ridurre le dispersioni idriche, di semplificare le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo nella realizzazione dei nuovi invasi, di pulire gli invasi esistenti,

Dalla disponibilità di acqua dipende la produzione degli alimenti, che sono alla base della nostra dieta mediterranea, molti dei quali vere e proprie eccellenze del *made in Italy*, dai formaggi ai salumi più conosciuti nel nostro Paese, ai vini, a tutto quello che è importante nel nostro panorama enogastronomico e nelle produzioni agroalimentari. Proprio per la volontà di preservare la qualità dei prodotti italiani, è stata autorizzata la sperimentazione in campo aperto delle tecniche di evoluzione assistita. L'emendamento, a prima firma del presidente della Commissione De Carlo, è stato approvato all'unanimità in Commissione, con la possibilità di aprire a questa norma, che consentirà alla nostra agricoltura di fare un grandissimo passo in avanti, sfruttando le tecniche di miglioramento genetico per produrre alimenti genuini e resistenti alla siccità e, in generale, alle condizioni meteorologiche avverse. Certo, avremmo voluto anche noi che non ci fosse stato imposto dal Governo il termine del 31 dicembre 2024. Ma, come ho detto direttamente alla senatrice a vita Cattaneo, vita Cattaneo, che stimo, questo termine non deve spaventarci, perché, come è stato detto in precedenza, abbiamo due provvedimenti e ne arriverà un terzo da esaminare congiuntamente in Commissione, per emanare, nell'arco di un anno, un provvedimento definitivo. Ci impegniamo inoltre affinché, nel caso in cui ci sia un ritardo da parte dell'altra Camera (non solo della nostra), ci sia la possibilità di prolungare questa azione, in modo tale che quelle cosiddette sperimentazioni, che dovrebbero durare tre anni, abbiano la possibilità di partire con un nostro impegno diretto e importante. L'inverno dal punto di vista climatologico ha fatto segnare una temperatura superiore di 1,21 gradi rispetto alla media storica, lasciando l'Italia per un lungo periodo nella morsa della siccità (non dimentichiamocelo), con danni stimati in 6 miliardi di euro per l'agricoltura. Per aiutare il settore ad affrontare questo difficile momento emergenziale, si è inoltre intervenuti sulla disciplina del deflusso ecologico, dando la possibilità, in presenza di prolungati fenomeni climatici avversi, quali proprio la siccità, di rimodulare le sperimentazioni su questo tema, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 6, della direttiva acque, riprese dalla legge n. 152 del 2006. evidente dunque che, subito dopo aver affrontato la fase emergenziale, con questo provvedimento dovremo agire con decisione sulla realizzazione di opere strutturali per garantire l'adeguata infrastrutturazione idrica al Paese. Non dimentichiamoci che lo stoccaggio dell'acqua piovana oggi è solo dell'11 per cento. I dati ci indicano che è una priorità assoluta l'assunzione di interventi volti a realizzare dei contenitori per aumentare la capacità di stoccaggio dell'acqua, ammodernando gli invasi esistenti e realizzandone di nuovi a livello territoriale, ma anche aziendale, come stabilito dal decreto. Diventa strategico per il Paese, accanto agli interventi emergenziali, dotarsi della realizzazione di un piano invasi (di piccoli e medi invasi), corredato da un realistico cronoprogramma e dal relativo piano finanziario. Questi contenitori artificiali, raccogliendo quantità importanti di acqua, consentiranno di poterle utilizzare, nei periodi di maggiore siccità, per usi agricoli, per uso civico, per uso industriale. Da ultimo, noi non possiamo non considerare gli impatti che ha avuto il cambiamento climatico sulle modifiche del ciclo idrogeologico nel nostro Paese. È per questo che dobbiamo guardare con particolare interesse al piano per il clima di prossima approvazione quale prioritario contributo alla realizzazione dell'obiettivo globale di adattamento ai cambiamenti climatici definiti dall'Accordo di Parigi. Questo diventa fondamentale. Signor Presidente, concludo ricordando a quest'Aula come negli ultimi anni abbiamo ricevuto importanti lezioni di vita, per noi impensabili. La pandemia ci ha insegnato quanto valore ha la prevenzione e la tutela della salute nel nostro Paese. La tragica guerra in corso quanto sia importante incentivare e tutelare la produzione energetica nel nostro Paese. La siccità prima e a seguire le piogge, alcune anche alluvionali, ci insegnano quanto siano importanti la tutela ed il contenimento dell'acqua, uniti alla preservazione dal rischio idrogeologico alluvionale dell'Italia.

Debbo ringraziare un po' meno il Governo, perché è accaduto, come le altre volte, che la maggior parte degli emendamenti e dei suggerimenti che sono venuti da maggioranza ed opposizione,

quanto questa problematica sia importante e significativa. Quindi, hanno visto che cosa c'è e soprattutto hanno visto che cosa non c'è

Se li hanno presentati, invece, in scienza e coscienza, allora forse il testo non era scritto bene e poteva essere migliorato in alcune parti. Noi abbiamo provato a farlo, purtroppo con esito insufficiente. In ultimo - fatemelo dire e mi rivolgo, sempre per il tramite della Presidenza, al Governo

siamo arrivati a discutere senza i pareri del MEF, tant'è vero che alcuni emendamenti della maggioranza sono stati ritirati per noia: perché a un certo punto, questi pareri non arrivavano ma dovevamo chiudere, quindi sono stati ritirati.

una gratitudine vera verso le rappresentanze sindacali, quelle di categoria, le professioni, l'associazionismo, che abbiamo ascoltato. Ci hanno davvero aiutato; per le poche correzioni e per i pochi miglioramenti che siamo stati in grado di fare, è stato determinante il loro contributo. Abbiamo discusso di quali politiche concrete mettere in campo contro il fenomeno della siccità e naturalmente lo abbiamo fatto - lo hanno ricordato anche coloro che sono intervenuti prima di me - nel mentre una parte di questo Paese era in una situazione

Discutiamo quindi di un provvedimento siccità e il Paese è alle prese con le alluvioni. In tanti lo hanno detto e lo voglio ribadire: non è una contraddizione, non è una alienazione dell'istituzione del Senato, perché stiamo parlando di due aspetti dello stesso fenomeno, che è quello del *caos* climatico. È vero, tale fenomeno può avere dei momenti di imprevedibile gravità, può generare eventi estremi e, nel momento in cui si presentano come estremi, travolgono tutto, qualunque tipo di prevenzione anche nella gestione del territorio. Tuttavia, che cosa è prevedibile? Che questo fenomeno tenderà a crescere, quindi ci saranno sempre più eventi estremi ed incontrollabili: è questa la sfida che abbiamo di fronte. Ne devono prendere atto anche il Governo e la maggioranza, che purtroppo in questi mesi nel dibattito pubblico, ma anche con le azioni politiche, ha dimostrato a più riprese di ignorare il problema dei cambiamenti climatici o addirittura di negarne l'esistenza, in ossequio a un approccio ideologico che si rivela negli effetti contro i territori e le comunità, oltre che contro la realtà e la scienza. Non partire da questo presupposto non ci consente una oggettiva analisi nel tempo presente e soprattutto nella prospettiva futura che siamo chiamati a interpretare, prima ancora che come legislatori, come cittadine e cittadini di questo Paese. Tanto più che, qualora servisse un ulteriore argomento a sostegno, la siccità ha fatto la sua parte anche nell'aggravare gli eventi calamitosi delle settimane passate, rendendo lo stato del terreno non in grado di ricevere e assorbire quantità di pioggia come quelle cadute. Serve dunque o, per meglio dire a questo punto della discussione, sarebbe servita un'iniziativa prima del Governo e poi del Parlamento diversa dal decreto-legge in discussione, per dare al Paese e ai territori una legislazione che affronti il fenomeno in modo strutturale, uscendo dalla precarietà delle soluzioni congiunturali. Così purtroppo non è stato: siamo di fronte a un provvedimento che, sebbene abbia visto interventi migliorativi, come ho detto, risulta lacunoso e non all'altezza del fenomeno. Possiamo dire senza timore di essere smentiti che si è persa un'occasione per dotare di norme e risorse le azioni di contrasto e prevenzione della siccità. Basterebbe ricordare come

sin dall'articolo 1, ma è rimasta la pregiudiziale e incomprensibile bocciatura dell'emendamento che avrebbero visto ragionevolmente la partecipazione del presidente dell'Associazione nazionale Comuni

quando bisogna affrontare questi momenti, bisogna dare protagonismo ai territori, non calare le scelte dall'alto. *(Applausi)*. Qualcuno qui dovrebbe insegnarcelo, visto che ne fa ampio vanto. Abbiamo insistito affinché si evitasse la previsione di un commissario autorizzato ad agire in deroga a tutte le norme ordinarie perché non serve certo un organo *legibus solutus* per affrontare il problema con un approccio che deve essere non verticistico; occorre piuttosto la condivisione è mancata la capacità del Governo e della maggioranza di concepire un provvedimento che mettesse al centro dell'attenzione la primaria esigenza di manutenere e ripristinare

Prima ho ricordato - e desidero ricordarlo anche adesso - che abbiamo cercato di ascoltare quello che è accaduto rispetto all'emendamento che abbiamo citato, frutto del confronto molto significativo Noi abbiamo provato ad essere liberi in questo confronto, quindi vi diciamo che il provvedimento in esame è del tutto insufficiente, ma continueremo a lavorare in Parlamento e nel Paese per insistere nel pretendere che chi governa e ha le responsabilità prenda a cuore l'idea che il Paese ha bisogno di una visione generale, di un provvedimento generale che sia capace di prevenire e non solo di inseguire i problemi.

doversi giustamente distinguere in Aula con evidenti dichiarazioni di voto poco rappresentative di ciò che è stato in realtà il lavoro in Commissione, che ha visto anche il loro contributo per migliorare il provvedimento. Questo, infatti, è un testo importante perché per la prima volta in Italia, quando si parla di acqua, non si parla solo di emergenza,

ma come si affrontano i problemi? Si affrontano con la demagogia, con l'ideologia, magari imbrattando sé stessi - poco male - o i monumenti per manifestare per il cambiamento climatico

lezioni che rimando al mittente, Presidente: chi ha il *record* mondiale di fiducie poste difficilmente può insegnare a noi cosa vuol dire svilire la discussione parlamentare, che è proprio quella che soprattutto in Commissione ci ha condotto ad approvare un numero di emendamenti

noi non prendiamo lezioni dagli amici del PD. Vi do un'altra grossa notizia che qualcuno pare aver dimenticato e cioè che tutte le operazioni che stiamo facendo le stiamo facendo perché abbiamo chiara e netta consapevolezza che sia in atto un cambiamento climatico

Scusate, colleghi, chiedo al senatore De Carlo di rivolgersi alla Presidenza e chiedo ai colleghi di lasciarlo parlare, come hanno lasciato parlare

si possano vedere dissalatori come in quei Paesi civilissimi che ne hanno già a iosa, ben sapendo che l'equilibrio ecosistemico va tutelato, ma lo sappiamo, perché è nel mezzo che sta sempre la bontà e la virtù e quindi il giusto equilibrio tra tutte tra tutte le risorse energetiche e idriche che mettiamo in campo. Finalmente è previsto l'utilizzo delle acque reflue anche in agricoltura. Per quanti anni abbiamo visto l'ideologia bloccare queste operazioni, che erano di fatto di buon senso? Finalmente abbiamo la possibilità di vedere bacini idroelettrici puliti, il cui costo non grava sulle spalle delle comunità locali. Ecco l'attenzione alle comunità locali: rendersi conto che, se è vero che i grandi gestori

adottando anche il potere sostitutivo nel caso di inerzia e quante volte dovremo utilizzarlo, quando non verranno spesi i fondi che si dovranno spendere. Lo faremo

produsse due spighe là dove se ne produceva una. Oggi possiamo mettere in campo la stessa rivoluzione, che vede protagonista l'agricoltore italiano, che oggi, signori, non è il grande inquinatore

il dissesto idrogeologico. Noi siamo convinti, signor Presidente, di aver contribuito con questo provvedimento a migliorare una situazione, mentre altri, per tanti anni, si sono semplicemente girati dall'altra parte, convinti o che il problema non ci fosse o che fosse talmente

che lascerei stare, se non fosse che ci sono di mezzo morti e famiglie in ginocchio. Non è affatto vero che ci sono stati soldi non spesi per la manutenzione

signor Presidente, ma ci tenevo a dire che sostenere che non sono stati spesi i soldi per l'idrovia padano-veneta non c'entra nulla con la tragedia alla quale siamo tutti vicini ed è inutile usare questa cosa per la polemica politica. Dico questo solamente perché rimanga gli atti di quest'Assemblea.

gli eventi climatici estremi e gli sconvolgimenti geopolitici di questi anni abbiano davvero reso palese che, per garantire la sostenibilità sociale, ambientale ed economica, oltre alla libertà sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, ci dobbiamo affidare all'innovazione e ai suoi strumenti scientifici e tecnologici. Le norme che consentiranno la sperimentazione in campo aperto di piante ottenute da nuove biotecnologie agrarie, che il Senato potrà oggi approvare, grazie alla meritoria attività dei senatori promotori e al voto unanime dei colleghi della Commissione, hanno un valore particolare, anche perché fanno sì che si affronti, sebbene parzialmente, il tabù della genetica in campo agrario, che da oltre vent'anni vede i nostri ricercatori pubblici prigionieri di un blocco scientificamente immotivato e dannoso per la società. Ecco, ho chiesto di parlare in dissenso dal Gruppo, ma questa circostanza eccezionale, di queste norme,

fanno sì che il mio voto, inizialmente orientato all'astensione, in dissenso dal Gruppo, a causa dei limiti culturali e politici che vedo in una norma che permette un'apertura selettiva solo ad alcune tecnologie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

La seduta è tolta